di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»,

XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci troviamo ora a discutere in Aula è stato approvato il mese scorso dalla Commissione igiene e sanità del Senato, dopo un lungo e travagliato percorso. Stiamo parlando del provvedimento in materia sanitaria, il quale è nato dall'esigenza di adottare ulteriori misure per garantire una maggiore funzionalità in diversi settori, in particolar modo quelli degli ordini e delle professioni sanitarie,

da esso, in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini in maniera più adeguata e più qualificata. Prima di discutere del provvedimento in questione, vorrei soffermarmi su un tema a me molto caro, per il quale ho condotto personalmente, e su diversi fronti, battaglie che mi hanno lasciato numerose cicatrici, ma sono fiero di averle combattute e per esse anche oggi in quest'Aula continuo a combattere. Cosa vuol dire sanità? Cosa intendiamo noi parlamentari, noi che abbiamo la responsabilità di agire in difesa del popolo italiano, quando parliamo di servizio sanitario? Il mio pensiero va immediatamente alla dignità dell'essere umano, fatto a immagine e somiglianza del suo Creatore, e ai diritti inviolabili che rendono la vita un bene prezioso; alla fratellanza in Cristo, che ci impone di non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, che ci consiglia di non esibire in pubblico la mano che dona speranza a chi è più sfortunato, che arriva persino a chiederci di pregare per i nostri peggiori nemici e per il loro bene; all'uguaglianza in suddetta dignità di tutte le persone e alla tutela del loro benessere, a prescindere da una condizione di Stato sociale, sesso, religione o etnia. Questo perché con tale provvedimento si vuole porre un nuovo riassetto della normativa vigente, che risale addirittura alla legge istitutiva degli Ordini del settembre del 1946, proponendo un sistema più aderente alle esigenze odierne e che possa assicurare la sua funzionalità nell'interesse dei cittadini. Per fare un esempio, da tempo esiste un problema serio, cui è urgente dare al più presto una risposta. Si tratta dell'irrigidimento delle attività e delle procedure della sperimentazione clinica, che non permette di adeguarsi in maniera rapida alle innovazioni sia tecniche che procedurali e che ha portato, inoltre, a una serie di criticità, come le diverse tipologie di contratto amministrativo per la sperimentazione, differenti da promotore a promotore e da amministrazione a amministrazione, o come il numero ridotto di centri di eccellenza in Italia. Il testo qui presentato prova a dare una risposta, prevedendo la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, seguito da un riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché nel rispetto degli standard internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione di Helsinki del 1964 e dalle sue successive revisioni. Sempre a proposito di sperimentazione clinica si prevede, inoltre, l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche nelle fasi dalla I alla IV, che prevedono la sperimentazione sulle persone; l'individuazione delle modalità per il sostegno all'attivazione e all'ottimizzazione dei centri dedicati agli studi, che devono fornire preliminari elementi per le valutazioni di sicurezza, sia su pazienti che su volontari, da condurre secondo i metodi della medicina di genere; l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti di interesse. Questo perché eventuali scoperte devono essere il frutto di una ricerca mirata al benessere della collettività, e non utilizzate per gli scopi economici di pochi industriali. Il testo propone un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, con appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme, all'interno del Servizio sanitario nazionale, e procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto in ostetricia, attraverso il ricorso a tecniche di anestesia loco-regionale, ma avremmo potuto prevedere, ad esempio, anche le tecniche di medicina complementare, quali l'agopuntura e la moxibustione. io stesso dimostrai l'efficacia dell'agopuntura in ginecologia e nell'ostetricia come alternativa al Policlinico universitario di Messina, nel reparto all'epoca diretto

della scuola argentina di Buenos Aires, negli Annali di agopuntura della scuola francese del professor Ngvyen Van Nghi, a Parigi e Marsiglia, e nella Scuola di medicina complementare a Colombo in Sri Lanka. Il punto focale del testo riguarda il riordino delle professioni sanitarie. Si tenta infatti di avviare una vera e propria rivoluzione nel settore attraverso la costituzione di nuovi albi, e il riconoscimento di nuove figure sanitarie. Vengono istituiti infatti ordini professionali, come quello per le professioni infermieristiche, le professioni di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ma non vengono delineati in modo chiaro percorsi formativi. Inoltre, nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti e dei biologi. È prevista poi l'istituzione e la definizione della professione dell'osteopata, la cui attività è subordinata all'iscrizione al relativo albo, possibile solo per chi è in possesso della laurea abilitante o dei titoli equipollenti. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono inserite le professioni di biologo e di psicologo. Per l'Ordine degli psicologi restano invariate le attuali norme organizzative, mentre l'Ordine dei biologi è inserito nell'albo dei chimici. Viene costituito l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri, con lo scopo di facilitare la circolazione di professionisti qualificati, con il vantaggio di avere una tecnologia efficace a supporto della diagnosi e della cura a costo sostenibile. La Commissione europea già da tempo preme per una ulteriore regolamentazione per quanto riguarda la professione dell'ingegnere biomedico, anche in considerazione del fatto che in Europa sono presenti oltre 25.000 imprese, soprattutto piccole e medie, che danno lavoro a ingegneri biomedici e ricercatori. È introdotto un inasprimento delle pene in caso di esercizio abusivo della professione sanitaria o di maltrattamenti e sono previste circostanze aggravanti per i reati commessi contro le persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. Riguardo al tema delle sostanze dopanti il provvedimento introduce una fattispecie di estensione, al farmacista, delle pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive considerate sostanze dopanti. L'estensione è prevista nei casi in cui il farmacista, in assenza della prescrizione medica, dispensi tali farmaci e sostanze per finalità diverse da quelle proprie, ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, con la previsione di pene da due a sei anni di reclusione e del pagamento di una multa da 5.164 a 77.468 euro. inoltre definite ulteriori modalità per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle attività ordinarie delle unità operative delle aziende del Sistema sanitario nazionale, con lo scopo di agevolare l'accesso dei giovani alla professione medica. Un ulteriore aspetto Il testo conferma il divieto di compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e farmacista. In altri termini, non potranno operare all'interno di una farmacia professionisti legittimati a prescrivere farmaci. Tutte le altre professioni, al contrario, sono ammesse. Nel caso in cui gli eredi siano tenuti a cedere la farmacia in mancanza di titoli universitari, il termine è stato innalzato da sei a quarantotto mesi. Un'ultima e non meno importante novità riguarda l'istituzione della professione di chiropratico e del relativo registro presso il Ministero della salute. Il rischio che nuove leggi, in un ambito così delicato come la sanità, possano portare a gravi ricadute sulla sicurezza e sull'affidabilità dell'organizzazione della salute pubblica è sempre presente ed è per questo necessaria un'attenta e precisa analisi al riguardo. Nei prossimi cinque anni si prevede che ci sarà una carenza di offerta sanitaria professionale dovuta allo sbilanciamento tra il numero di medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale che andranno in pensione ed il numero di nuovi laureati in medicina e chirurgia e in veterinaria. Ciò richiede, quindi, un ripensamento più adeguato ed efficiente del nostro sistema sanitario, sempre più martoriato dai continui tagli alla spesa pubblica, tenendo presente anche il recente calo dell'aspettativa

laddove è necessario e giusto rielaborare specializzazione e competenze in base alle continue modifiche della società, in termini di necessità del paziente e progressi della ricerca, non dobbiamo dimenticarci che una buona metà dell'intera professione è rappresentata dal rapporto con gli ammalati. Ippocrate ci insegna che bisogna entrare nelle case per portarvi sollievo e lo stesso San Luca, da medico e fratello in Cristo, fu l'unico ad accompagnare Paolo nei durissimi giorni del carcere, fino all'atroce supplizio che gli si parava dinnanzi. Anche nel Levitico, in particolare nei passi relativi alla cura della lebbra Il malato veniva condotto dal sacerdote, responsabile del benessere spirituale, fisico e psicologico del proprio popolo, al fine di tenerlo in osservazione, senza affrettarsi ad emettere una prognosi negativa, per sbarazzarsene prima possibile. Al contrario, nelle nostre università la semeiotica medica non viene più considerata materia obbligatoria ed è stata tolta dal piano di studi. Eppure la Bibbia ci insegna che nessun malato, soprattutto cronico, va abbandonato al proprio destino, tanto meno eliminato in funzione di un'aspettativa di vita basata su meri calcoli statistici, che troppo spesso non coincide con la reale morte. Lo stesso Gesù ci insegna che la vita è sacra e lo fa proprio in quell'uliveto in cui verrà arrestato per essere portato al Tempio, in catene, come un criminale: ammonisce San Pietro, che stava cercando di difenderlo con la forza e la violenza, ricordandogli che «chi di spada ferisce, di spada perisce». Una dimostrazione di compassione evangelica vera e radicale, che in Italia si svolge nel quotidiano di una corsia ospedaliera costantemente sotto organico, dove mancano posti letto, medicinali, addirittura garze o siringhe, e dove i miracoli, nonostante la buona volontà degli ultimi angeli che vi lavorano, purtroppo non avvengono più a causa della necessità di fare cassa. Non posso fare a meno di ricordare in quest'Assemblea le mie continue battaglie contro le *lobby* del farmaco e lo stato di precarietà lavorativa in cui versano persone che dovrebbero salvarci la vita. ripeto: riorganizzare o modernizzare è giusto, ma la cosa importante è tenere sempre a mente che la sofferenza non può attendere ed è mio dovere di cittadino, di medico, di politico e di cristiano non voltarle mai le spalle, lavandomi le mani e la coscienza con la consapevole bugia di un futuro più organizzato e moderno, Concludo, signor Presidente, ribadendo una verità innegabile: in campo medico organizzazione e modernità non devono significare produttività e profitto,

Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, la Presidente della Commissione igiene e sanità, che è anche relatrice del provvedimento, mi ha cortesemente - e anche correttamente - chiesto di sedere ai banchi della Commissione. Credo infatti sia giusto che la politica esca dal perimetro asfittico di una contesa che molto spesso ci allontana dal conseguimento degli obiettivi e dia - anche plasticamente se possibile - alla comunità un senso di unità, allorquando ricorrano le condizioni e quando vi sia una ragionevole convergenza di vedute, di sensibilità e di valutazioni, che portano al conseguimento di un medesimo obiettivo. Ebbene, credo che il faticoso lavoro compiuto in Commissione igiene

rispetto all'accoglimento delle posizioni, delle obiezioni, delle valutazioni e delle perplessità, che si sono sostanziate non solo in sede di discussione generale, ma anche attraverso l'elaborazione e la presentazione di emendamenti, molti dei quali sono stati approvati in Commissione e alcuni dei quali approdano all'Assemblea per un ulteriore e più collegiale approfondimento. Ebbene, credo che quel sistema di lavoro sia la traccia più interessante, come metodo: parte dalla 12a Commissione il segno di una politica che recupera il proprio ruolo, la propria funzione e probabilmente, attraverso questo recupero, si candida anche a riparare quel corto circuito che si è determinato nel tempo tra la piazza e il palazzo. Entriamo ora nello specifico. percorso è stato lungo, tormentato, accidentato, tribolato, non privo di*scoop* dell'ultimo momento, come ricorderà la mia amica e collega Laura Bianconi, relativamente ai disegni di legge attinenti parte degli argomenti che formano oggetto di questo disegno di legge cosiddetto Lorenzin

accadeva di tutto. Credo che questa volta il «di tutto» non accadrà, se non la conferma di un lavoro approfondito, circostanziato, puntuale, che anche grazie alla presenza del Governo si è potuto svolgere

assolutamente necessario, coerente con i tempi, misurato, equilibrato, utile per una serie di motivi. Entriamo nel merito con un con un percorso molto rapido sugli aspetti che, a mio sommesso avviso, rappresentano i punti caratterizzanti di questo disegno di legge.

ed esteso a materie sì contigue ma eccessivamente rilevanti, al punto tale da non poter essere affrontate tutte

perché attengono ad argomenti rilevantissimi. Ne cito solo due: la sicurezza alimentare e la sicurezza veterinaria, che rappresentano punti di forza nell'azione legislativa che sorregge un impianto normativo funzionale alle esigenze di una sanità più sicura e al conseguimento di maggiori e migliori obiettivi di tutela della salute. L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di riordino delle norme sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Io sono stato un fervido censore delle deleghe al Governo; lo sono stato perché molto spesso sono state deleghe indefinite, larghe e ampie, che hanno portato, poi, non poche sorprese. Questa è una delega "palettata", come si dice in gergo, ben circoscritta, dove la funzione del Governo è individuata in modo puntuale e preciso. Credo che essa vada nella direzione di semplificare, per un certo verso, le norme in materia di sperimentazione, ma sempre garantendo - anzi, più e meglio di quanto non accadesse prima - i requisiti necessari affinché quella sperimentazione conduca fuori da conflitti di interesse. Attraverso una migliore declinazione dei principi di trasparenza, emergono le finalità di una sperimentazione che, naturalmente, deve deve servire primariamente, in modo deciso ed evidente, al conseguimento di nuovi sistemi di terapia che concordino con i progressi delle scienze scienze mediche e farmaceutiche. Il riferimento, nell'articolo 1, alle modalità di conduzione dei sistemi di sperimentazione

dal vocabolario del legislatore con una declinazione concreta, che non è così aleatoria o sospesa nell'auspicio e nei desideri ma si attua

Finalmente si arriva ad introdurre nei livelli essenziali di assistenza il parto indolore: una conquista di civiltà.

talvolta convergenti e talvolta profondamente divergenti e difformi rispetto alla disciplina degli ordini professionali.

agli ordini professionali delle funzioni sanitarie - la loro funzione pubblicistica, abbiamo preso questa decisione nella consapevolezza che il punto di criticità di questa analisi non stava nelle strozzature ideologiche - ordini sì, ordini no - ma nella constatazione che la normativa di riferimento degli ordini professionali è datata 1946. Colleghe e colleghi, 70 anni fa veniva approvato il decreto luogotenenziale n. 233 del Capo provvisorio dello Stato. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 1946. È cambiato un mondo e noi abbiamo preteso che in questi 70 anni gli ordini continuassero a declinare le proprie funzioni pubblicistiche ispirandosi a

un'azione degli ordini professionali insufficiente e talora addirittura una funzione che ha tradito le sue iniziali prerogative. Credo tuttavia che quelle prerogative siano state recuperate in modo preciso. Sapete perché, colleghe e colleghi? Per un semplice motivo. Nel testo di legge è scritto in modo chiaro ed inequivocabile che gli ordini «sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari

che, nella declinazione verticale dei compiti, dallo Stato fin giù al territorio, garantisce di più e meglio, nel comparto che stiamo esaminando, le esigenze del cittadino. Attraverso l'attività di vigilanza e di controllo e i compiti che nell'articolo 3 vengono dettagliati puntualmente, in relazione ai percorsi formativi e alla verifica

è un fatto assolutamente importante. A questo si aggiungono anche aspetti di non poco conto, che hanno rappresentato un'ombra - per così dire - sulla funzione e sull'autonomia degli ordini professionali. L'azione disciplinare, fino ad oggi concentrata nello stesso organo rappresentativo della professione, il consiglio direttivo, da domani, con l'approvazione di questo disegno

una funzione disciplinare che si attenua, sino ad annullarsi, per motivazioni spinte dalla logica della corporazione, che ha il sopravvento sulla funzione pubblicistica. Tutto questo non accadrà più, perché vi è una separazione fra la funzione giudicante e la funzione istruttoria; mi sembra cosa assolutamente non da poco. Non mi attardo sugli aspetti di maggiore rilievo, che ancora potrei evidenziare in relazione all'articolo 3. 3. Mi limito a ricordare che, rispetto al tribolato percorso dell'Atto Senato n. 154 nella precedente legislatura, che prevedeva l'istituzione di ben 18 albi

I collegi degli infermieri e delle ostetriche vengono trasformati in ordini. Vorrei riferire un fatto semantico. Nel 1946 c'era la distinzione solo per i percorsi formativi diversi: i primi avevano un percorso che non prevedeva la laurea, gli altri (medici, farmacisti e veterinari) avevano invece la laurea. Oggi tutti hanno la laurea e tutti sono giustamente classificati in ordini. inoltre la trasformazione del collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie e tecniche della riabilitazione e della prevenzione. Quindi all'interno di questo Ordine confluisce la professione di assistente sanitario. Credo sia un ammodernamento che disciplina, puntualizza e precisa, senza tuttavia essere pletorico rispetto alla rispetto alla proliferazione di nuovi ordini.

Liquido subito il dibattito che ha conosciuto anche fuori da quest'Assemblea toni grevi e insufficientemente giustificati La Commissione 14a, nell'esprimere il proprio parere in merito al disegno di legge, dice espressamente che le figure professionali di osteopata, agopuntore e chiropratico, di cui si prevede la regolamentazione, sono già previste in alcuni Paesi europei con un livello di qualificazione che varia da tre a quattro anni di formazione universitaria, a più più di quattro anni. Anche qui, sgomberiamo il campo dagli equivoci; non ci sono attenzioni e premure per alcuni e distrazioni per altri. C'è la necessità di dare garanzie al cittadino perché il disegno di legge ha un elemento centrale nel suo obiettivo: dare garanzia di efficacia ed efficienza al cittadino, tutelandolo sotto il profilo della salute pubblica. Non è possibile che ci siano attività professionali che non siano disciplinate e riconosciute perché - attenzione, mi rivolgo anche a chi oggi ottiene questo traguardo - ottenere il riconoscimento vuol dire assumere delle responsabilità

all'atteso e necessario recepimento dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, che sostanzialmente prevede la possibilità di svolgimento nella farmacia di attività che non siano quelle del medico, da quella di prescrizione, perché il rischio comparaggio è in agguato. Tuttavia, alle professioni sanitarie non dotate di potestà legislativa si consente la possibilità di svolgimento

finestra") *(PD)*. Egregio Presidente, signore senatrici, signori senatori, intervengo sul disegno di legge su cui stiamo riflettendo e ragionando dopo aver ascoltato con molta attenzione gli interventi che mi hanno preceduto e che hanno evidenziato tutte le caratteristiche di questo disegno

Questo provvedimento riporta norme che si riferiscono ad aree tematiche diverse, ancorché collegate da un filo rosso conduttore: tutte ineriscono ai molteplici ambiti che caratterizzano la salute e la sanità del nostro Paese. La mia riflessione e il sostegno fortemente convinto all'intero disegno di legge sono comunque orientati ai numerosi articoli che trattano il tema delle professioni sanitarie. Finalmente, dopo un lasso temporale ben più che decennale, sì è giunti, da una parte, al riordino e alla novellazione delle norme che riguardano i modelli e le strutture di valutazione, validazione e rappresentanza delle professioni sanitarie; dall'altra, a dare pari riconoscibilità e dignità anche a numerose professioni sanitarie già regolamentate con specifici profili delineati e formalizzati con appositi decreti dal Ministero della salute e che, da oltre un ventennio, si formano in università attraverso percorsi di laurea triennale, quinquennale e *master* di primo e secondo livello. Queste ultime professioni sanitarie, peraltro, sono ancora inopinatamente mantenute prive di propri albi professionali, oppure con albi professionali inseriti nella struttura collegio, piuttosto che in quella di ordine. Il riordino e la novellazione delle norme inerenti alle professioni sanitarie e i modelli e le strutture di loro validazione, valutazione e rappresentanza, possono compiutamente essere definite come un ulteriore passo in avanti non tanto e non solo per gli oltre 1,2 milioni di professionisti sanitari operativi nel nostro Paese, quanto per i cittadini italiani ed europei che fruiscono delle loro prestazioni professionali e del loro impegno assistenziale. La tanto attesa riforma ordinistica in sanità si lascia alle spalle, finalmente, un percorso tortuoso e accidentato fatto di *stop and go*, di speranze e acerbe delusioni rese ancora più incomprensibili per l'acclarata evidenza di quanto il previgente e attuale impianto ordinistico avesse bisogno di un'ampia ridefinizione nei contenuti, nelle forme di partecipazione al voto, nei modelli di *governance* interna (sia a livello locale che regionale e nazionale), nei rapporti con le diverse istituzioni e con i propri professionisti, nei contatti e nella rete di rapporti con la collettività e con i singoli cittadini, che diventano attori protagonisti nella gestione, attraverso la mediazione, dell'eventuale e sperabilmente raro contenzioso.

che con il provvedimento in argomento, approvato all'unanimità dalla 12a Commissione del Senato, avvicinano ancora di più il nostro Paese all'Unione europea, in quanto facilitano la realizzazione dei disposti di due recenti decreti legislativi.

comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle etichette mediche emesse in un altro Stato membro; nonché al decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva n. 55 del 2013 dell'Unione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del 2005 e 1024 del 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno IMI. In entrambe le direttive, integralmente recepite dal nostro Paese con i succitati decreti legislativi, viene dato e riconosciuto un ruolo significativo agli ordini professionali sanitari e alle funzioni che tali enti dovranno svolgere a favore dei cittadini proprio per la loro funzione di enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dell'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Il decreto legislativo n. 38 del 2014, all'articolo 5, dispone che i pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a informazioni su vigilanza e valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria e su quali di loro sono soggetti a standard e orientamenti per le opzioni terapeutiche su fatture, prezzi ed onorari, su *status* di autorizzazione dei professionisti, sulla loro copertura assicurativa, responsabilità professionale o altri mezzi di tutela personale e collettiva. Sempre il decreto legislativo n. 38 del 2014, all'articolo 7, dispone che gli attivandi punti di contatto per l'assistenza sanitaria transfrontaliera forniscano anche informazioni sui prestatori di assistenza sanitaria e sul loro diritto ad esercitare o sulle restrizioni all'esercizio professionale. Nel decreto legislativo di cui trattasi, si afferma infine, all'articolo 11, che l'Italia si impegna affinché le informazioni sul diritto di esercizio professionale dei professionisti sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel territorio nazionale siano, su richiesta, messi a deposizione degli altri Stati dell'Unione europea.

Ancora, il decreto legislativo n. 15 del 2016 definisce, all'articolo 4, come professione regolamentata l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti locali pubblici,

mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale di indicate professioni sanitarie. A questo punto è ben evidente, dunque, il ruolo fondamentale che gli ordini professionali sanitari dovranno svolgere a favore dei cittadini-pazienti per quanto attiene ai dati, alle informazioni, alle competenze dei loro iscritti e alla garanzia di professionalità di cui questi ultimi devono essere in possesso. È altrettanto ben evidente che l'uniformità applicativa delle norme ordinistiche a tutte le professioni sanitarie fornirà e darà maggiori garanzie ai cittadini tutti, oltre che ai professionisti iscritti. Credo sia importante sottolineare, a conclusione di questo intervento, che gli ordini professionali sono emanazione della volontà dello Stato e dei professionisti di darsi delle regole chiare, trasparenti e lineari per un esercizio professionale di alta qualità e di garanzia nei confronti dei loro assistiti, e che tali organismi sono e saranno completamente autofinanziati dai professionisti stessi. Un ulteriore contributo dato dagli stessi al buon andamento del sistema salute nella sua globalità, senza ulteriori oneri per i cittadini e per le istituzioni. Quello degli ordini e dei professionisti iscritti agli albi è, quindi, un impegno a favore dell'intera collettività sociale, che potrà contare su solidi, attenti

Credo sia la dimostrazione - ove mai ce ne fosse bisogno - della necessità e dell'opportunità che il Governo non usi, come spesso e volentieri fa, un'azione muscolare di prendere o lasciare, soprattutto proponendo provvedimenti cosiddetti *omnibus*.

alcuni parti del provvedimento, non perché non meritevoli di attenzione, ma in quanto necessitavano assolutamente di un approfondito esame a parte. Parlo della sicurezza alimentare e della sicurezza veterinaria, tanto richiamate nei giorni precedenti relativamente alla salvaguardia dei famosi prodotti *made in Italy*, ma importanti soprattutto in relazione alla garanzia di una sicurezza alimentare nei confronti dei cittadini.

dal Governo. È opportuno, visto che si parla tanto di Parlamento (e la Commissione ha dato dimostrazione delle sue possibilità), che anche l'Assemblea e il Parlamento si riapproprino delle loro funzioni. Mi auguro che il passaggio

di tutte le persone interessate, e soprattutto (e questo credo sia l'aspetto più importante dal punto di vista politico), malgrado sollecitazioni a volte anche eccessive da parte di - chiamiamole si è appropriata della propria autonomia decisionale e, dopo aver sentito tutti, ha deciso nell'interesse più generale e non nell'interesse particolare. Questo credo sia l'aspetto politico fondamentale e più importante, utile nel prossimo futuro

Il provvedimento certamente non è il migliore in assoluto. Ricordavo prima che partiamo da alcuni provvedimenti del 1946, ed è evidente che il mondo è cambiato anche in materia sanitaria e nelle professioni; quindi bisogna riconoscere quali sono le novità, le opportunità e soprattutto le garanzie per quanto riguarda i cittadini e in particolare i pazienti, perché sappiano a chi rivolgersi con garanzie da parte del potere dello Stato. Questo è il punto fondamentale.

fatto nell'interesse più generale, come il provvedimento in Commissione ha saputo fare. Ringrazio i componenti della Commissione

Signor Presidente, questo disegno di legge contiene tematiche complesse e diversificate che, come ci ricordava il senatore Zuffada, abbiamo esaminato in Commissione sanità in modo molto analitico, approfondito, anche attraverso un percorso partecipato e l'audizione di molti soggetti interessati, che ci ha portato alla formulazione di disposizioni molto attese come il riordino delle professioni (sulle quali non entrerò perché ci sono colleghi che lo hanno fatto e lo faranno meglio di me), o di principi come l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica, l'assenza di conflitti di interesse e l'indipendenza dello sperimentatore. Inoltre, l'articolo 6 prevede l'aggravante per i reati contro le persone presso strutture sanitarie e sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali. È insopportabile quello che troppe volte ci viene restituito dalla cronaca. Sono negli occhi e nei cuori di tutti le tragiche immagini di anziani maltrattati in strutture sanitarie Questo articolo 6 è davvero di grande importanza. Mi soffermerò invece sulle questioni che più mi stanno a cuore come la medicina di genere. Per lungo tempo, la differenza tra uomini e donne è stata ignorata o considerata un fattore secondario nello sviluppo di nuove soluzioni farmacologiche e nell'individuazione di trattamenti e forme di prevenzione delle patologie. Il pregiudizio secondo cui il corpo della donna è uguale a quello dell'uomo ha pervaso la medicina ed è duro a morire. Ancora oggi tale pregiudizio inficia gran parte della ricerca medica e farmaceutica. I risultati ottenuti nell'uomo vengono acriticamente trasposti nella donna, secondo un errore metodologico grave che ha portato, non dobbiamo dimenticarlo, a due grandi tragedie: quella del talidomide, che ha avuto come esito la nascita di bambini focomelici, questione ancora in discussione in Parlamento, in attesa di una soluzione giusta e dignitosa che ci auguriamo possa arrivare presto, o quella del dietilstilbestrolo, un estrogeno che veniva somministrato durante la gravidanza e che poteva causare complicanze e neoplasie nelle bambine. Adottare in campo sanitario e farmaceutico una prospettiva di genere vuol dire ridisegnare i trattamenti, includere espliciti obiettivi di genere attraverso programmi di prevenzione, formazione del personale medico, parità di accesso ai servizi sanitari, significa cambiare le basi della ricerca e la sperimentazione clinica prevedendo che ad essa partecipino con un'adeguata presenza sia donne che uomini. L'evoluzione della ricerca e della formazione medica in questo campo è molto recente e piuttosto lenta. Per questa ragione è particolarmente importante che la 12a Commissione abbia integrato il disegno di legge originario prevedendo uno specifico riferimento alla medicina di genere nella delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica. L'articolo 1, come modificato dalla Commissione, infatti, nel delineare i principi e i criteri direttivi della delega precisa, alla lettera *c)*, che l'individuazione

È ormai diffusa la convinzione che sia necessario un approfondimento scientifico del fatto che donne e uomini presentano, nell'arco della loro esistenza, patologie differenti o differenti sintomi di una stessa patologia. La conoscenza delle differenze di genere favorisce, infatti, una maggiore appropriatezza Nonostante esistano significative differenze che influenzano diversamente il metabolismo dei farmaci nelle donne, rispetto agli uomini, una buona parte delle molecole, come ad esempio alcuni psicofarmaci, non è stata sperimentata sulla popolazione Salto alcuni argomenti e mi riservo di consegnare la relazione, ma voglio ricordare una cosa molto importante. Questa legge prende atto di tali novità e, con l'articolo 2, imprime un'accelerazione nel campo delicatissimo del dolore connesso al parto, un campo storicamente carico di significati simbolici. L'articolo 2 prevede, infatti, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza riguardo alle prestazioni di controllo

che l'aggiornamento dei LEA deve tenere conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all'interno del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento al nostro esame segna, un primo importante passo avanti nell'affermazione dei diritti delle donne, nell'affermazione della differenza femminile come valore anche nel campo fondamentale della prevenzione, della malattia e della cura. La diffusione dell'analgesia porterà inoltre sicuramente ad una contrazione dei parti cesarei, riportandolo su valori medi nazionali,

stato di salute di un'intera popolazione e rappresenta la cartina di tornasole delle pari opportunità in un settore rilevante, anche da un punto di vista costituzionale, qual è quello della salute.

connessi** Gentili colleghe e colleghi, innanzitutto vorrei esprimere un sincero ringraziamento alla relatrice per l'ottimo e paziente lavoro svolto in Commissione in tanti mesi di ascolto dei numerosi professionisti e associazioni del settore sanitario. Era assolutamente necessario dare ordine, trasparenza, sicurezza sia agli operatori che ai pazienti, soprattutto dopo l'introduzione, negli ultimi 20 anni circa, delle innovative professioni sanitarie. C'era, inoltre, assoluta necessità di un riordino complessivo della disciplina degli ordini professionali. C'era bisogno inoltre, proprio per il rispetto che si deve alle persone che hanno necessità di cure, che ci fosse un aumento delle pene per coloro che esercitano abusivamente la professione: serve rassicurare i pazienti ma anche i tanti, tantissimi professionisti che ogni giorno svolgono con dedizione e abnegazione il proprio lavoro, facendo in modo che la nostra sanità, e lo possiamo dire con orgoglio, possa ancora essere tra le migliori al mondo. Per questo la previsione di pene che possono essere aumentate da un terzo fino alla metà di quanto previsto dall'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo. abusivo. Altro importante segnale di grande attenzione alle persone più fragili, con la modifica dell'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti, è quello di punire più severamente coloro che commettono reati a danno di persone che sono ricoverate presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali. Pensiamo a quante volte ci affliggiamo o ci siamo rattristati per notizie di cronaca che riguardano ragazzi e ragazze disabili accolti in centri residenziali o semiresidenziali; o anziani accolti

Come è stato sottolineato poc'anzi dalla senatrice Granaiola, ma mi piace ritornare sulla questione toccandone altri aspetti, una delle più significative innovazioni introdotte in Commissione durante l'esame del disegno di legge, su cui vorrei soffermare la mia attenzione, è il riferimento esplicito, all'articolo 1,

La garanzia di un approccio metodologico in materia di sperimentazione clinica fondato sulla medicina di genere rappresenta un passo fondamentale compiuto nell'universo sanitario e volto a organizzare approcci terapeutici differenziati che sappiano tener conto delle differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne. In tal modo sarà possibile orientare percorsi specifici per le donne, anche in relazione al settore della ricerca medica. La pubblicazione del Quaderno del Ministero della salute del 22 aprile scorso si inserisce proprio nell'ottica di sviluppare un contesto di riferimento appropriato volto a dare il rilievo che merita alla dimensione di genere. Le differenze biologiche e socio-culturali tra gli uomini e le donne influenzano l'incidenza delle malattie, la presentazione clinica e gli effetti delle terapie, rappresentando un punto di rilievo interessante. Dunque, la prospettiva di genere, come già evidenziato negli anni '90 dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, è da includere all'interno di una scelta politica, soprattutto riguardo alla salute fisica e mentale, dato che la ricerca in campo medico è stata fondata prevalentemente sugli uomini. Il genere, in relazione alle più recenti politiche sanitarie europee, è stato ritenuto dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un elemento essenziale per la promozione della salute, nella direzione dello sviluppo di approcci terapeutici differenziati

il fatto che il testo sia stato licenziato all'unanimità è la migliore espressione di una sinergia e di una sintonia che, al di là delle diverse appartenenze politiche, è stata raggiunta. Va dato atto alla presidente De Biasi di questa questa ritrovata unità, ma non è che questo provvedimento risolva i problemi, che sono ancora molteplici, affinché il Servizio sanitario nazionale possa essere ancora più efficiente e soprattutto possa essere compatibile con le risorse finanziarie assegnate. Non voglio sembrare un bastian contrario, ma continuo a ripetere che tutti gli sprechi e gli sperperi che la gestione statale della sanità determina

È invece noto che questo aspetto, al di là dei personali convincimenti, viene trascurato, quasi che lo Stato, depositario di un'etica superiore dei fini, potesse continuare impunemente a sprecare e a sperperare, senza che questo possa essere oggetto di censura o senza che questo vada a gravare sulla parte meno abbiente della popolazione. Come dimenticare la stagione dei *ticket*? Come dimenticare il fatto che la sanità è la terza voce di spesa

approntare nuovi protocolli terapeutici per patologie che oggi non sono adeguatamente sostenute dal Sistema sanitario nazionale.

pertanto la riflessione che vorrei pacatamente fare in quest'Aula è che ci si dovrebbe domandare perché il nostro Sistema sanitario,

di un sistema che continua a fare debiti e che vede alcune Regioni (alcune più buone, altre meno buone)

per la parte non statale, alla determinazione di contratti, che, caro Sottosegretario, sono stati utilizzati in alcune Regioni per sviare surrettiziamente l'utenza obbligata a servirsi solo delle strutture pubbliche.

continuiamo a lamentarci ed è una gara di tipo solidaristico tra chi è più buono e chi lo è meno. Io forse sembro meno buono perché metto il coltello nella piaga, perché vivo sulla mia pelle di professionista, da trentacinque anni, questa sperequazione. Dico questo non per tutelare interessi diffusi di una categoria, che pure sono legittimi. Attenzione.

cui nel Centro-Nord si è obbligati ad utilizzare le strutture statali (ovviamente obblighiamo chi non ha la tasca piena, perché chi ha la tasca piena se ne frega dell'obbligo). in un sistema sanitario in cui lo Stato divide il Fondo sanitario non tenendo conto della diversa produzione di ricchezza delle Regioni. Un cittadino lombardo spende 1.860 euro, che corrispondono alla quota capitaria, e ci rimette altri 550 euro di tasca propria.

per cui abbiamo le Regioni canaglia, che sono quelle che devono friggere il pesce con l'acqua, e le Regioni virtuose, la cui popolazione può sopperire con propri mezzi e con proprie risorse al *deficit* del sistema.

C'è un errore materiale, che pregherei il Governo di rimuovere e che credo sia sfuggito anche alla Commissione, nelle

invece di scrivere il «Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi» è stato scritto il «Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi», che è cosa diversa.

Dovrebbe essere previsto e specificato, anche se si tratta di una legge delega, che così come accade per le altre professioni sanitarie, anche i chiropratici debbano conseguire una laurea magistrale e credo anche un corso di specializzazione, per tutte le altre professioni che entrano nella dimensione sanitaria è previsto il massimo della formazione e della specializzazione. Mi avvio dunque alla conclusione: la salute è trascurata, perché quando uno ce l'ha, non se ne cura, e inizia a preoccuparsene quando viene meno. Credo che il nostro compito sarebbe quello di avere cura della salute di tutti, con un sistema basato sull'efficienza, sulla produttività, sulla competenza e sul merito. Ebbene, serve un sistema flessibile, che garantisca la libera scelta del cittadino a quelle strutture pubbliche che erogano prestazioni di maggiore complessità e di migliore qualità. Abbiamo già introdotto, legge finanziaria da poco approvata, il criterio per cui tutti gli ospedali vengano parametrati con pagamento a prestazioni secondo delle tariffe. Estendiamo questo criterio ovunque,

quello - diciamolo - è l'emblema del politico di turno, che esibisce l'ospedale zonale come il raggiungimento di uno scopo. Quelli sono ospedali inutili e pericolosi

nonostante le barelle fuori dalla porta, l'ospedale, pagato a DRG, chiuderebbe il 30 giugno. Immaginate qual è lo spreco e lo sperpero nel più grande ospedale del Mezzogiorno. Continuando a pagarlo a piè di lista, il Cardarelli produce 100 milioni di euro di debito all'anno, chiunque vada a gestire la Regione Campania, e quei 100 milioni sono sottratti alla povera gente. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, va premesso che nel testo del provvedimento approvato dalla 12a Commissione troviamo indubbiamente novità positive e, come qualcuno ha ricordato, anche lungamente attese, dal 1946. Per esempio, l'aver reso operante il concetto di medicina di genere, ormai patrimonio universale della comunità scientifica, l'aver introdotto norme sulla sperimentazione clinica e sulle modalità di revisione dei LEA. E, a proposito dei primi due articoli, vale la pena di sottolineare il giusto spirito di semplificazione che percorre la materia trattata. Quanto alle professioni sanitarie, sono indubbiamente positivi sia la trasformazione dei Collegi in Ordini, che il riconoscimento del ruolo professionale, con l'istituzione di Ordini e Albi, di alcune figure sanitarie che ricoprono un ruolo sempre più importante nella tutela della salute dei cittadini: mi riferisco ai biologi, agli psicologi, ai chimici e ai fisici e al passaggio di queste quattro professioni sotto la vigilanza del Ministero della salute. Ma anche l'istituzione di nuove professioni, come quella di chiropratico e quella di osteopata, e l'accorpamento nell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, di professioni sanitarie tecniche, come quelle della prevenzione e riabilitazione, che non hanno ancora Albi professionali pur essendo regolamentate. Infine, l'istituzione, presso l'Ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici è sicuramente un fatto importante. Tali misure vanno senz'altro a tutelare i professionisti, ma soprattutto, ed è quello che ci deve interessare di più, i cittadini, che fruiscono delle loro prestazioni in maniera certa e sicura. Ritengo, poi, sia un passo avanti fondamentale aver riassorbito nel testo che stiamo discutendo il disegno di legge n. 693 che io ho presentato all'inizio di questa legislatura. Tale proposta è volta a modificare l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, così da permettere esplicitamente all'interno della farmacia l'esercizio delle altre professioni sanitarie, con l'ovvia eccezione di quelle abilitate alla prescrizione, come ha ricordato qualche collega prima di me: medico, odontoiatra e veterinario. si allinea questa materia alle necessità del modello della farmacia dei servizi introdotto dalla legge n. 69 del 2009, a tutto vantaggio del servizio che potremo offrire ai cittadini. Sono anche stati apportati miglioramenti della normativa che renderanno più agile e meno onerosa la vita degli Ordini professionali, come la previsione che i consigli direttivi durino in carica quattro anni.

non possiamo tacere qualche zona d'ombra e non possiamo nascondere che questa distinzione poteva essere meglio articolata ed essere accompagnata da una maggiore graduazione delle sanzioni. Da sempre, infatti, gli Ordini professionali si trovano nell'impossibilità legale di commisurare, come ho detto, con la giusta gradualità, le sanzioni alle violazioni commesse e questo è sicuramente un elemento che rende più difficile contrastare i comportamenti illeciti. Infine, vorrei fare un rilievo che credo sia il più importante e che nasce dalla riaffermazione contenuta nel testo, per me essenziale che gli Ordini delle professioni sanitarie sono enti pubblici non economici e organi sussidiari dello Stato, ovviamente

Il punto è che il testo conferma la costituzione degli Ordini professionali nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province vigenti al 31 dicembre 2012. Il mio pensiero, oggi, in queste ore, in questi giorni, va dunque alla riforma costituzionale che sarà oggetto di *referendum* confermativo in autunno. Infatti, proprio alla luce delle considerazioni svolte, si aprono due scenari:

la sanità rimane una competenza regionale, per cui mi chiedo, proprio per l'esperienza di questi anni, come una rappresentanza professionale provinciale potrà rapportarsi in maniera efficace e coerente nella rappresentanza regionale cui fa riferimento. è un po' l'incompiuta, il nodo ancora da sciogliere: di fronte ad una riforma costituzionale importante, rimane un'asimmetria che, nell'uno e nell'altro caso, non potrà che essere affrontata al più presto, per rendere davvero gli Ordini più moderni e capaci di rispondere alla sfida che vogliono portare avanti.

Una innovazione che parte dal Capo I e dall'articolo 1, che tratta il tema della sperimentazione clinica dei medicinali e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, e lo dico a partire dalla medicina di genere, che è un approccio diverso ed innovativo, indispensabile per superare le disuguaglianze di salute. Questo è uno dei temi più rilevanti, Questo è uno dei temi più rilevanti, perché la promozione della ricerca e della sperimentazione differenziata in base al genere è necessaria per affrontare le disuguaglianze di salute e per garantire la parità di trattamenti e di accesso alle cure, nonché l'appropriatezza delle cure stesse. Per lungo tempo la differenza tra uomini e donne è stata considerata un fattore secondario, sia nello sviluppo di nuove soluzioni farmacologiche che nella individuazione di forme di prevenzione e trattamento delle patologie. Lo dimostra, fra l'altro, una tradizione di studi registrativi effettuati prevalentemente su pazienti maschi e l'effetto di questa minore presenza di donne nei *trial* è quello di terapie che non sempre e non pienamente sono adeguate alle esigenze della salute e cura delle donne. Invece, la medicina di genere è uno dei modi migliori, ad esempio, per dare concretezza al concetto di centralità del paziente, sia nella ricerca e nella messa a punto di trattamenti efficaci ed innovativi, sia per la personalizzazione delle cure. La dimensione di genere nella salute è una necessità di metodo e di analisi ma diviene anche uno strumento di governo del sistema. Dunque, riconoscere la differenza di genere diventa essenziale per delineare i programmi, organizzare l'offerta di servizi e garantire l'appropriatezza. Siamo tutti impegnati, in questo tempo, a sostenere e rafforzare la qualità del Sistema sanitario nazionale e sappiamo bene che per dare concretezza a questo obiettivo servono politiche di appropriatezza

per l'attivazione e l'ottimizzazione dei centri clinici da condurre con approccio metodologico di medicina di genere, nonché, come ho detto, la necessità che la sperimentazione clinica sui medicinali, debba essere svolta su una adeguata rappresentatività di genere. Inoltre, si prevede anche una cosa importante che riguarda la formazione: per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati, si stabilisce che debba includersi la farmacologia di genere. Altrettanto importante è l'articolo 2, quello sull'aggiornamento dei LEA, che stabilisce in modo chiaro che essi debbano tener conto delle specifiche esigenze della medicina di genere, prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme nel Sistema sanitario nazionale. Ho parlato di grande innovazione e mi riferisco ancora al Capo I, parlando dell'importanza della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle normative in materia di sperimentazione clinica di farmaci innovativi, sostanzialmente per rafforzare la ricerca clinica. Rilevante è il fatto che andiamo a potenziare esattamente la sperimentazione clinica, il cui obiettivo è quello di migliorare, potenziare e dare trasparenza ed efficacia alla ricerca clinica, attraverso scelte significative come la definizione di procedure di valutazione e di autorizzazione nella sperimentazione clinica, nonché l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati, così come l'individuazione di modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e garantire l'assenza di conflitti di interesse,

che riguarda la revisione normativa relativa agli studi clinici senza scopi di lucro. Tra l'altro, questa è una richiesta fortemente sostenuta da tutte le associazioni del *non profit*. È davvero di grande rilievo la promozione e il sostegno della ricerca indipendente e dell'iniziativa formativa che

garantire l'uso delle risorse già a disposizione e semplificare le procedure amministrative, comprese le assicurazioni, per sperimentazioni, così come indicato dal regolamento europeo n. 536 del 2014, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento. Termino sottolineando anch'io l'importanza dell'articolo 6, che, con riferimento all'articolo 61 del codice penale, definisce come circostanze aggravanti l'aver compiuto reati in danno di persone in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali. Questo è un primo importante segnale, una risposta importante ai troppi episodi che si verificano, così come ci dimostrano le cronache, nei confronti di anziani non autosufficienti o di disabili, persone che hanno necessità di una cura attenta, amorevole e di grande professionalità. Io so che certo non basta intervenire sulla pena: dovremmo affrontare in modo celere e più generale la questione a partire dalla prevenzione e dalla formazione del personale piuttosto che dai controlli. Ma intanto questo provvedimento si fa carico del pezzetto di propria competenza. Ritengo che anche questo sia uno degli elementi che hanno testimoniato, intorno a questo provvedimento, una grande unità e una grande discussione, appassionata e competente, in Commissione e mi sembra che anche in Aula ci sia lo stesso sostegno. L'auspicio è che questo disegno di legge venga approvato rapidamente e che altrettanto rapidamente la Camera possa recepirlo.

È vero che questo disegno di legge contiene una delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, oltre che in materia di aggiornamento dei LEA, di riordino delle professioni sanitarie e, infine, sulla dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Partendo dalla sperimentazione clinica, in Commissione sanità si è posta la nostra attenzione rispetto agli *standard* internazionali per l'etica della ricerca medica sugli esseri umani, con la definizione delle procedure per la verifica dell'indipendenza e dell'imparzialità degli sperimentatori e, infine, per far sì che in questa sperimentazione ci sia un'adeguata rappresentanza di genere. Sono tutte cose che sembrano scontate a questo punto, ma che hanno avuto un'ampia discussione in Commissione. Detto questo, credo che, siccome si tratta di una legge delega, dobbiamo anche dire cosa avremmo potuto fare e cosa ancora siamo in grado di fare per poter migliorare questo nostro lavoro. Dato che l'articolo 2 introduce il riferimento alla medicina di genere, che rivolge una particolare attenzione ad una fase importante della vita della donna come il parto, spererei che con il tempo un'analoga attenzione venga data anche alle fasi che precedono il parto e in proposito mi viene mente una cosa sulla quale ho discusso più volte anche in Aula, che è l'interruzione volontaria di gravidanza. di gravidanza. Secondo me sarebbe giusto affrontare in maniera consapevole il problema dell'obiezione di coscienza, cioè il famoso articolo 9 della legge n. Che ci siano reparti di ginecologia dove si arriva al 90 per cento di obiettori è scandaloso, visto che il servizio pubblico deve garantire l'interruzione volontaria di gravidanza a tutte le donne che fanno questa scelta che ricordo - è sempre una scelta dolorosa e non viene fatta così, tanto per piacere. Non dobbiamo nemmeno, come è successo in quest'Aula, nasconderci dietro i numeri statistici.

Ritengo che dovremmo fare in maniera che in ogni reparto di ginecologia sia garantito questo servizio e per questo i non obiettori dovrebbero essere il 70 per cento e non viceversa. Spero che il Parlamento si attivi per risolvere questo

È una scelta importante quella di inserire nei LEA le procedure per il controllo del dolore, sia nel travaglio che nel parto, anche attraverso il ricorso all'anestesia locoregionale. Quello che manca, a mio avviso, è che non riusciamo ad inserire nei LEA le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita. Vengono erogati dal Sistema sanitario nazionale i farmaci che sono necessari alla procreazione medicalmente assistita e non inseriamo le

che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 40 del 2004 nella parte in cui vieta le tecniche di fecondazione eterologhe, avremo un aumento di questa tecnica. da una notizia di oggi, ci dice che una coppia su tre paga il trattamento di tasca propria e la cifra si aggira oltre i 5.200 euro. I centri pubblici sono pochi e lunghe sono le liste di attesa. Teniamo presente che la percentuale di gravidanze su donne trattate è attualmente al 22 3, recante il riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie. finalmente modificare questa struttura e di farlo in maniera così precisa e puntuale. Diciamo anche, però, che uno dei problemi principali degli Ordini sanitari, ma in pratica di tutti gli Ordini professionali, è quello della democrazia interna e della trasparenza degli atti. La trasparenza non è un fatto che riguarda solamente gli iscritti agli Ordini, ma anche i cittadini, in quanto le decisioni di questi Ordini hanno sicuramente ricadute certe sulla società. Non solo; dalle modalità di elezione dei vertici sia a livello provinciale che nazionale, derivano tutta una serie di cariche (previdenziali, tipo quelle per le pensioni, o per la gestione dei beni immobiliari) e di consulenza presso organismi istituzionali interni al Sistema sanitario nazionale. Aumentare il livello di democrazia interno agli Ordini è dunque, secondo me, prioritario. Sino ad ora gli accordi tra le entità di maggior peso all'interno degli Ordini hanno determinato eletti e politiche senza che all'interno delle assemblee elettive sia stato possibile avere una vera e propria opposizione riconosciuta dal voto degli iscritti. Sarebbe quindi necessario che le elezioni avvenissero nel riconoscimento di liste contrapposte. Posso dire che questo tema riguarda da vicino l'Ordine dei medici-chirurghi: pensate che a Firenze, su 7.000 iscritti, vanno a votare soltanto 1.500 medici, perché sanno che tanto quella sarà la lista vincitrice e sanno anche che non ci sarà una vera democrazia all'interno dell'Ordine, senza che all'interno delle assemblee elettive sia stato possibile avere una vera opposizione riconosciuta per il voto degli iscritti. Su questa base, ho proposto un emendamento con cui chiedo

Inoltre, proprio a protezione da eventuali conflitti di interesse sarebbe opportuno che per gli organismi provinciali e nazionali la durata in carica sia di quattro anni, per non più di due mandati consecutivi, imponendo di fatto un ricambio automatico delle rappresentanze: fino ad oggi, infatti, ci sono stati Presidenti che hanno raggiunto e superato i dieci anni di mandato. Altrettanto importante, secondo me, è la questione del peso che ogni singolo ordine ha sull'elezione di organismi nazionali. Ad oggi i vertici di ogni categoria professionale in campo sanitario sono determinati da un numero ristretto di Ordini provinciali, che hanno un elevato numero di voti a disposizione e possono eleggere un rappresentante ogni 200 iscritti.

È necessario salvaguardare il principio per cui un Ordine con un numero maggiore di iscritti ha un peso più grande, ma non a scapito della democrazia. Per questo motivo, in Commissione abbiamo innalzato l'elezione di un rappresentante ad ogni 500 iscritti. un passo avanti, ma ritengo che si dovrebbe arrivare ad un rappresentante ogni 2.000 iscritti, lasciando comunque gli Ordini con meno di 2.000 iscritti la possibilità di eleggere ugualmente un loro rappresentante. Questo renderebbe più democratica la rappresentatività.

i Collegi delle ostetriche divengono Ordini della professione di ostetrica. All'articolo 4 viene istituita e definita la professione di osteopata; all'articolo 5 l'ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo, all'articolo 6 l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici. clinici. A fronte di tutto questo, credo sia venuto il momento di non ignorare più la figura del dottore in scienze motorie. So di andare contro corrente rispetto al parere della Commissione, ma tale figura, con le sue diverse specializzazioni, è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione e della salute in diversi ambiti, senza alcun riconoscimento professionale da parte dello Stato. Pensiamo non solo all'educazione motoria a scuola, che a mio avviso deve raggiungere i livelli dei sistemi scolastici del Nord Europa, ma anche ai centri *fitness*, alle palestre, alle strutture sanitarie, alle associazioni sportive. Quando si parla di salute non possiamo affidarci a personale non qualificato e mentre è vero che posso controllare in quale palestra va mio figlio a cinque o sei anni, non posso assolutamente sapere e controllare dove va mio figlio che ne ha 25, che a volte torna a casa imbottito di anabolizzanti semplicemente perché è finito in una palestra dove la figura professionale non esiste affatto. Si tratta di un problema serio perché, soprattutto nelle prime fasce di età. L'educazione motoria svolta in maniera scorretta influisce gravemente sullo sviluppo e sulla salute del bambino, e di conseguenza dell'adulto. Inoltre - lo abbiamo detto tutti - ogni euro speso in prevenzione tramite una corretta educazione motoria consente di risparmiare oltre quattro euro di spese sanitarie.

è stata riconosciuta come malattia, in Italia le persone in sovrappeso sono oltre 21 milioni; questo comporta una diminuzione della speranza di vita da cinque a La prevalenza è tra i 55 e i 74 anni, mentre la percentuali di bambini obesi è del 9,8, con percentuali più alte nelle Regioni del Centro e del Sud. È evidente ed è chiaramente fondamentale che, nonostante il fatto che i laureati in scienze motorie impiegati nel mercato del lavoro continuino a vantare un tasso di occupazione superiore alla media, uno dei punti più critici è rappresentato dall'elevatissima quota di lavoro sommerso. Inoltre, chi non lavora in nero è spesso costretto a firmare contratti atipici e precari, pur lavorando come dipendente a tempo pieno. La percentuale di laureati con contratto a tempo indeterminato è infatti molto bassa. A complicare ulteriormente la situazione - e lo abbiamo visto in Commissione sanità poi il problema della condivisione degli spazi con i fisioterapisti: una storica guerriglia fatta di invasioni di campo e gelosie professionali; laureati in scienze motorie da una parte, fisioterapisti dall'altra. Credo sia arrivato il momento di sanare in maniera corretta la disparità di trattamento di questi professionisti. Se, infatti, al dottore in scienze motorie è negata la possibilità di operare come fisioterapista come ritengo giustissimo - a quest'ultimo è concesso di operare in ambiti propri del laureato in scienze motorie. È questo quello che fanno tanti operatori, spesso con competenze tecniche acquisite - è vero ma privi della qualificazione universitaria indispensabile per interventi che riguardano la salute, la prevenzione, i processi educativi, l'equilibrio psicofisico. Un luogo comune è che la laurea in scienze motorie sia relativamente facile da acquisire. Molte persone pensano che la maggior parte degli studenti passi il proprio tempo all'università praticando le più svariate discipline sportive, divertendosi e dedicando soltanto una minima parte allo studio

recita che: il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree: didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili; tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline; manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive. In parole spicciole, e facendo un po' di interpretazione su quanto scritto dal legislatore, il laureato in scienze motorie avrebbe competenze (non esclusive) e possibilità di lavoro in ambito scolastico, nelle palestre o centri *fitness*, nell'intervento rieducativo, nella preparazione atletica e nell'ambito manageriale. Questa interpretazione è resa necessaria dal fatto che nel decreto legislativo citato non si parla di che cosa il laureato in scienze motorie faccia o possa fare, ma in realtà solo delle conoscenze che dovrebbe possedere. Distinzione che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto, poiché vi è differenza fra il possedere delle conoscenze ed esserne poi l'esecutore unico, deputato a mettere in pratica le stesse. Da qui si viene a creare l'equivoco di fondo del laureato in scienze motorie, custode di conoscenze messe poi in pratica da tutti. Di certo è che in questo settore specifico sembra essere davvero il momento di trovare soluzioni concrete. L'inserimento e la pratica dell'educazione fisica all'interno delle scuole non deve trattarsi più di un mero ideale, ma di un fatto concreto, vista l'importanza fondamentale che il movimento riveste per l'armonico sviluppo psico-corporeo nell'età evolutiva. Anche il progressivo inserimento del laureato all'interno del mondo universitario renderebbe gli insegnamenti sicuramente più interessanti e le docenze più credibili. Non è possibile che un insegnamento in didattica dell'attività motoria possa essere svolto da laureati in lettere o filosofia, con tutto il rispetto che nutro per questi ultimi. A noi A noi legislatori spetta il compito di fare leggi giuste, in maniera che, in questo caso, in campo sanitario, la differenza, quella vera, la facciano la preparazione, la competenza, la voglia. Per questo motivo chiedo, e credo che sia giunto il momento, di istituire anche l'albo dei laureati in scienze motorie.

ha visto il suo esordio più di vent'anni fa. Parliamo di oltre 800.000 operatori per i quali l'*iter* del percorso di organizzazione delle professioni sanitarie è iniziato con la legge n. 502 del 1992, proseguendo con la legge n. 251 del 2000, fino alla legge n. 43 del 2006. Quest'ultima ebbe il grande merito di prevedere una disciplina organica all'interno della quale era prevista una delega al Governo per l'istituzione di ordini professionali nel settore sanitario. Queste importanti innovazioni non hanno mai visto la luce. La delega di fatto è rimasta inattuata per scadenza dei termini. È indubbio che le questioni sanitarie rappresentino un elemento centrale nell'organizzazione sanitaria nazionale, in una sanità che che è profondamente cambiata. Oggi parliamo di diritto alla salute, del primariato della prevenzione, di un sistema solidale e universalistico, ed è indubbio quindi che i professionisti siano veramente l'asse portante, gli attori principali di tutto ciò. Purtroppo provvedimenti non adeguati o disattesi hanno creato nel tempo disparità e commistioni tra disposizioni di principio e norme di dettaglio. L'assenza di un filo conduttore legislativo moderno, al passo con i tempi, ha reso difficile rispondere alle sempre maggiori richieste di professionalità provenienti dal cittadino utente. Ben sappiamo che esistono ragioni moderne che si appoggiano su problemi antichi e sappiamo anche che i tempi e gli attori sono profondamente cambiati. Ma quello che con tenacia e coraggio tentiamo di fare in questo provvedimento è proprio di non nasconderlo, e di affrontarlo con equilibrio. Appare evidente che l'impianto ordinistico in sanità ha bisogno di un profondo adeguamento normativo nei contenuti, nella modalità di partecipazione, nei rapporti con i cittadini. Non possiamo non legiferare, non possiamo più tergiversare, non possiamo lasciare al libero mercato o all'anarchia la soluzione di tali problema. A tal proposito, a chi critica questo provvedimento perché in controtendenza con la necessità di liberalizzare, ricordiamo che neanche la Commissione europea si è mai sognata di seguire questo disegno per le professioni sanitarie, capendo molto bene che la materia di cui parliamo è estremamente delicata e complessa. di un atto di giustizia, di riconoscimento, di promozione della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e dei percorsi formativi per essere riconosciuti come tali; ma è anche ma è anche una legge a tutela dei cittadini in un comparto colpito pesantemente da un odioso e grave abusivismo professionale. Credo che ognuno di noi su questo testo avrà ricevuto centinaia di *e-mail* - lei, signora poche a favore, molte in disaccordo. Molte di queste *e-mail* erano volte a tutelare la propria professionalità rivendicando percorsi e discorsi che appartengono al passato. A tutti gli operatori e al mondo politico, che ha lavorato con impegno su questo provvedimento, desidero rivolgere due ultime considerazioni. il tempo è passato, le situazioni nel tempo si sono consolidate e si sono affacciate altre prospettive. Il difficile equilibrio trovato dentro questo provvedimento può sicuramente scontentare qualcuno e far gioire altri, ma è un equilibrio e bisogna porre sulla bilancia questo risultato possibile rispetto a un non possibile risultato. E, credetemi, non ho alcuna certezza che questa volta potremo scrivere la parola fine. La seconda considerazione è che anche su questo tema abbiamo visto la politica sostenere tesi discordanti, a volte anche con posizioni fantasiose, ma in politica dobbiamo riconoscere che vige la norma di grande saggezza che i nostri Padri costituenti ci hanno tramandato e che troppo spesso dimentichiamo: non si legifera contro qualcuno, ma si cerca di costruire, facendo del proprio meglio, una legge che possa migliorare la vita di tutti.

si affaccia definitivamente la medicina di genere. Lo voglio ricordare in questa Aula perché la prima volta che il Parlamento si è occupato di medicina genere è stato in questo Senato, nel lontano 2003, attraverso una mozione *bipartisan*. Era una materia allora sconosciuta. D'altronde, era una materia molto giovane. Era nata come idea nel 1976 da una cardiologa statunitense che si era si era scocciata di vedere risultati diagnostici e terapeutici distinti tra uomini e donne: gli uomini venivano curati meglio per i farmaci dati rispetto alle donne. Da allora nacque un movimento. Stiamo parlando di pochi anni. Eppure, questo movimento ha preso fiato grazie al nostro interessamento. Lo dobbiamo dire: questo Senato se n'è fatto parte attiva. Non so se il presidente Calderoli, che nel 2003 era vice presidente, presiedesse quella seduta l'Aula. Mi sembra di ricordare questo.

I collegi accademici, i convegni e le altre mozioni hanno fatto sì che oggi diventasse patrimonio comune e finalmente lo troviamo scritto a chiare lettere come un diritto sancito all'interno di un provvedimento. È anche per questo che

tra audizioni, discussione generale, emendamenti e approvazione. È stato oggetto di analisi in 53 sedute della Commissione sanità. Questo serve a capire come sia stato profondo lo studio su questo provvedimento. È iniziato, come è stato ben spiegato, con 26 articoli, ne sono stati stralciati 16 e ne sono stati aggiunti 4. Vorrei leggere il titolo di alcuni articoli stralciati come, per esempio, la delega al Governo sul riordino degli enti vigilati, in materia di sicurezza degli alimenti, in materia di navi frigo finalizzate alla prevenzione del

Ciò evidenzia come il Governo sia ormai abituato a costruire provvedimenti disorganici che raccolgono decine di criticità che tentano di risolvere senza una visione organica e complessiva. Così, capita sovente che la toppa sia peggio del buco. È molto interessante l'introduzione dello specifico riferimento alla medicina di genere. Credo che nella sperimentazione tutte le variabili debbano essere prese in considerazione e non solo la medicina di genere, ma anche, ad esempio, l'età. Ricordo l'insegnamento dei miei professori di pediatria, che mi dicevano che un bambino non è un uomo piccolo, ma che ha una sua psicologia, fisiologia e patologia diverse dall'adulto. È comunque molto importante che un argomento così complesso come la sperimentazione clinica venga finalmente disciplinata, anche in riferimento al nuovo regolamento europeo e alla Dichiarazione di Helsinki. Una considerazione anche sull'articolo 2, che aggiorna i LEA, e sul contenimento del dolore nella fase del travaglio del parto.

recante il riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie. Sul fatto che gli Ordini andassero rinnovati e rivisti siamo tutti perfettamente d'accordo. In questo provvedimento si disciplinano alcuni

articolo organizza gli Ordini secondo un assetto strutturale molto simile al vigente. Nasce una struttura verticistica abbastanza impositiva, che permette agli iscritti un potere decisionale quantomeno nelle scelte organizzative, considerato anche che devono pagarsele. Affrontiamo ora alcune criticità che voglio qui sottolineare. Considerare Considerare che siano le Federazioni nazionali a chiedere la riunificazione e lo sdoppiamento di circoscrizioni non appare funzionale. Difficilmente gli Ordini propongono l'accorpamento nonostante non siano in grado di funzionare. Pertanto, in tal senso sarebbe più opportuno che l'accorpamento fosse disposto dal Ministero. Sarebbe più opportuno comunque un'articolazione quantomeno regionale, in armonia con la struttura regionale del Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che già oggi alcuni Ordini

Riconoscere che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali siano enti pubblici non economici contrasta con la reiterata volontà di sottrarsi all'applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e a tutte le norme pubblicistiche tipiche della pubblica amministrazione, come l'anticorruzione e la trasparenza. Anche Anche l'autonomia professionale finanziaria così ampia non si concilia con la natura di ente pubblico non economico e di organo sussidiario dello Stato volta a tutelare

La verifica dei titoli abilitanti all'esercizio professionale è di facile reperimento, essendo un titolo che si consegue all'università ed autocertificabile. Anche la pubblicità integrale degli elenchi è necessaria per non comprimere la concorrenza e la reale possibilità di scelta tra tutti gli operatori professionali di un albo e per specifiche competenze. La pubblicità integrale di tali elenchi consentirebbe di accertare il reale numero degli iscritti all'albo, la loro funzione nella società, il gettito derivante dall'introito delle quote obbligatorie di iscrizione. di iscrizione. Assegnare agli ordini la programmazione dei fabbisogni di professionisti, ovvero del loro numero è assai discutibile ed è giustificata dal fatto che questi enti dovrebbero avere il polso della situazione occupazionale dei loro iscritti. Sulla base di ciò, prima dell'inizio dell'anno accademico, dovrebbero fornire al Ministero della salute il numero degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea di pertinenza. Ciò non avviene, però, perché gli Ordini nella maggior parte dei casi non conoscono la reale situazione occupazionale dei propri iscritti.

sovrastimato per soddisfare le esigenze degli atenei e giustificare l'apertura o il mantenimento di corsi di laurea con pochi studenti, da cui usciranno professionisti che, data l'attuale crisi occupazionale, resteranno, con una discreta probabilità, senza lavoro. Gli Ordini non hanno interesse a diminuire il numero degli iscrivibili adeguandolo alle esigenze professionali. Inoltre, il fatto di rivestire un ruolo nel mondo accademico e, contemporaneamente, una carica elettiva all'interno di un Ordine garantisce un futuro bacino di voti da quegli studenti che saranno un giorno

la formazione è un valore costituzionalmente garantito ed è libera. Nel caso dei professionisti della salute è stato introdotto invece l'obbligo di acquisire formazione cosiddetta ECM erogata da *provider*, autorizzati dal Ministero della salute tramite una Commissione nazionale ECM di cui peraltro fanno parte i rappresentanti del mondo ordinistico.Vale la pena sottolineare che anche taluni ordini, direttamente o per tramite di fondazioni da essi costituite e poco trasparenti, sono accreditati come *provider* di formazione ECM. Anche la gestione dell'attività disciplinare, così come descritta alla lettera *i)* del comma 2 dell'articolo 1 appare ridondante, poco funzionale e più attenta a tutelare gli interessi corporativi. Anche in questo caso c'è un conflitto d'interessi macroscopico laddove soggetti eletti e/o eleggibili sono anche soggetti giudicanti e soggetti legiferanti. Tra l'altro, la funzione giudicante è notoriamente discrezionale e non è prevista una precisa corrispondenza tra infrazione e sanzione. Inoltre molti professionisti sono dipendenti pubblici già sottoposti a norme disciplinari delle aziende di appartenenza e devono essere sottoposti anche al regime disciplinare ordinistico. Anche il fatto che il collegio dei revisori dei conti debba essere elettivo, nell'ambito di professioni che poco hanno a che fare con competenze tecnico-amministrative, appare assai discutibile. È assurdo che nel terzo millennio i revisori dei conti di un ente pubblico non economico non siano revisori contabili, come previsto dalle norme sul controllo interno di ogni pubblica amministrazione e come previsto, tra l'altro, dalle recenti norme istitutive dell'elenco dei revisori contabili presso il MEF. Si mantiene quindi l'assurda previsione che medici, infermieri e ostetriche eletti siano revisori contabili di una pubblica amministrazione.

e questo crea il perpetuarsi di una serie di persone che restano in carica per moltissimo tempo. Tra i compiti assegnati al consiglio direttivo vi è per esempio «la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari». Il parere sulla liquidazione degli onorari non ha ragione di esistere a fronte dell'abolizione delle tariffe.

che non sono aperti al pubblico e che non garantiscono la funzione di tutela collettiva a loro demandata. Infatti i rari casi di scioglimento degli Ordini avvengono solo per contese politiche elettorali e non perché notoriamente non funzionanti. un altro punto del provvedimento si prevede che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo (questa previsione è priva di ogni logica, sia nel caso dei pubblici dipendenti, sia nel caso in cui l'abilitazione professionale è data da un titolo universitario); avere la residenza e/o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. Questa è una limitazione chiaramente anacronistica rispetto all'evoluzione dettata dall'informatica e dalla rete, che rende ormai pleonastica l'esistenza di albi correlati alla residenza o al domicilio. Inoltre non si concilia con il libero esercizio della professione sia sul territorio nazionale che su quello europeo, talché è evidente che la stessa struttura territoriale degli Ordini non è più rispondente alla funzione degli Ordini stessi né alla libera circolazione dei professionisti. Anche il fatto di essere cancellato dall'albo professionale per morosità è un atto da valutare con attenzione: oltre a rilevare il carattere paratributario del contributo di iscrizione, nonché il potere impositivo degli ordini, si può in tal modo inibire l'esercizio di una professione. Oggi tutti i professionisti, terminati gli studi universitari, hanno la necessità di iscriversi e quindi pagare una quota e nel frattempo non lavorano o lavorano in maniera così precaria che non raggiungono neanche la sopravvivenza.

si sarebbero dovuti inserire nell'istituendo Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica delle prevenzioni sanitarie e tecniche e della riabilitazione e prevenzione tutti gli altri albi di professionisti che ci siamo dimenticati, dal logopedista, al podologo, all'ortottista (ce ne sono veramente tantissimi).

Il sistema già prevede l'eventuale istituzionalizzazione di nuove figure professionali attraverso il meccanismo previsto dalla legge n. 43 del 2006, che possiamo così sintetizzare: recepimento di direttive comunitarie, ovvero per iniziativa di Stato e Regioni; accordo della Conferenza Stato-Regioni che definisce il titolo professionale e l'ambito di attività; parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità allargato agli esperti del Ministero della salute, delle Regioni e degli Ordini professionali; funzioni che non devono essere parcellizzate e sovrapporsi alle funzioni delle professioni già esistenti. Detto questo, appare evidente che l'istituzionalizzazione della professione di osteopata ha un suo percorso e, alla prima occasione di riconoscimento di nuove figure professionali, il legislatore non solo smentisce sé stesso, ma percorre due strade, una per gli osteopati e un'altra per i chiropratici. Dunque, l'osteopata viene riconosciuto per legge ordinaria senza pareri tecnici, senza un precedente fabbisogno riconosciuto dai piani sanitari e senza neanche la necessità di dover dare un ambito giuridico a figure che operano nel Servizio sanitario nazionale, in quanto totalmente assente dalle strutture. Curiosamente, la norma rimane in vigore, ma non vale per questa occasione. Il collega Romani ha già evidenziato la criticità tra queste figure e la laurea in scienze motorie e non intendo oltre. Avremmo voluto capire come intendete organizzare i corsi universitari di laurea triennale, comuni alle molte professioni con specializzazione con un *master* di uno o due anni successivi

inoltre messo mano alle scuole professionali rivolte agli studenti *post* licenza media, che creano delle professioni il cui ruolo, a questo punto, non è del tutto chiaro.

di un provvedimento che è di interesse di molte persone e di tantissimi professionisti della salute.

anche l'esame degli emendamenti, che sono pochi e facilmente affrontabili.

l'immagine che diamo all'esterno non sia certamente piacevole, diciamo così.

da vent'anni sta aspettando gran parte delle norme contenute nel provvedimento in esame, certamente non capisce né questa melina, né questo ostruzionismo,

riforma costituzionale, verrà consegnato ad altri stili e ad altre persone, lo dobbiamo anche a noi stessi e al lavoro che normalmente facciamo con estremo impegno e serietà nelle Commissioni competenti. Questo è vero in modo particolare nella Commissione sanità che, signora Presidente, mi pregio di poter dire, lavora veramente molto seriamente e con passione. Ripeto la polemica di ieri: probabilmente, se uno dei colleghi che, anche quest'oggi, ha chiesto la sospensione venisse a lavorare in Commissione sanità non darebbe sponda a richieste pretestuose come questa*. (Applausi

le motivazioni che inducono molti senatori, anche in termini di ampia rappresentanza politica, ad esprimere valutazioni tendenzialmente positive e di convergenza sul lavoro che è stato fatto.

buona parte delle norme in esso contenute furono già approvate dalla Camera dei deputati cinque anni fa. Ne cito una sola, quella che assegna un percorso giuridico e scientifico alla ricerca.

talché sono i magistrati, poi, a stabilire se si debba irrogare una determinata terapia, per quanto aleatoria e non scientificamente validata. validata. Il bicameralismo ci ha portato, dopo cinque anni, a riproporre le cose che all'unanimità approvammo alla Camera e che non si poterono approvare al Senato voi ritenete opportuno, rispetto a un problema di carattere sociale, scientifico e culturale di così vasta portata, come quello della disciplina del percorso scientifico sulla sperimentazione clinica di farmaci o di terapie innovative, venire a perdere tempo su queste questioni? Fate ostruzionismo sulla bollinatura dei prosciutti della Val Brembana, ma lasciate perdere queste che sono cose serie e vanno oltre la strumentalità del gioco politico! Noi dobbiamo procedere perché dobbiamo recuperare cinque anni di tempo per milioni e milioni di persone malate che attendono, probabilmente, che la scienza dica una parola in loro soccorso, tale da ascoltare la verità scientifica e non la verità degli azzeccagarbugli che ogni tanto si parano sulla scena della pubblica opinione, proponendo cure miracolose per malattie rare. si abbia un minimo di senso di responsabilità relativamente all'argomento che si intende rimandare. Ci sono mille modi di fare ostruzionismo e mille modi di perdere tempo ma non è certo questo l'argomento sul quale esercitare

siete ritornati tutti in Aula e quindi, convinti di questo, ridiamo dignità all'Aula e ritiriamo la richiesta di chiusura anticipata

chiedere la fiducia al Parlamento, nel caso specifico al Senato, dovrebbero al Senato dare fiducia. Questo ha dimostrato il metodo con il quale abbiamo

Tant'è vero che molti emendamenti presentati anche da Forza Italia, che mi onoro di rappresentare in Commissione, sono stati accettati e fanno oggi parte del testo presentato.

che questa legge, che è appunto una legge di delega al Governo, non debba subire ritardi. Non può subirne, signor sottosegretario De Filippo, anche perché alcuni argomenti che abbiamo trattato in Commissione hanno rilevanza di carattere europeo e potrebbero,

noi riteniamo che, se il Governo dovesse proporre ulteriori tagli alla salute, bene farebbe a rinunciare ad un sistema olistico ed universale.

Ricordo che, allo stato attuale, la normativa che regola questa professione è contenuta nell'articolo 12 del regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle

professionisti, che pagano le tasse e che difendono posti di lavoro per migliaia e migliaia di persone. L'Italia

che vedono nella professione degli ottici optometristi la possibilità di creare mercato, di creare posti di lavoro e di pagare le tasse.

Questa è una forte ingiustizia; l'attività degli ottici professionisti viene riconosciuta in tutte le Nazioni europee. Bene, rivolgo un'ulteriore appello al Governo e alla Commissione igiene e sanità: fate giustizia, fate giustizia! La delusione non ha nulla a che vedere con il riconoscimento delle altre professioni, ma è legata alla constatazione che ci sono delle forti *lobby* che bloccano lo sviluppo e la crescita di questa professione. Si tratta di un'ottusa sordità o di una cecità selettiva; tale incapacità di comprendere l'evoluzione di una categoria

in ottica e optometria. In questo Parlamento invece non è data dignità a questa professione. Ebbene, faccio un ulteriore appello al Sottosegretario e alla Commissione: ritengo che ci siano le condizioni perché si possa trovare una soluzione per riconoscere questo diritto.

signor Sottosegretario, presidente De Biasi, colleghi, oggi andiamo a trattare un tema che non solo risponde a criteri di grande attualità e di grande richiesta, ma anche ad una sintonia

e, in particolare, per quanto riguarda l'aggiornamento degli stessi LEA con inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase di travaglio e di parto. È un tema che rappresenta una testimonianza tangibile di una civiltà assistenziale, di un *modus agendi* da tanto tempo atteso e da tantissime donne richiesto in tutto il territorio nazionale e non a macchia di leopardo come si caratterizza l'assistenza in sala parto solo e soltanto in alcune zone d'Italia. A me sembra, signora Presidente, che questa tematica crei una declinazione di apertura da una riflessione squisitamente in ambito bioetico e della biomedicina in un ambito più correttamente di ordine biopolitico e - oserei dire - di ordine "biolegislativo". non nell'ottica della biopolitica, come veniva richiamato dal suo mentore Michel Foucault, vale a dire come un dominio della politica e dell'arte politica sul corpo, sulla vita della donna e sul corpo in genere, ma come una nuova forma paradigmatica in cui il rispetto e la dignità dell'essere donna, dell'essere persona nel momento del travaglio, possa avere un suo riconoscimento nobile, un'intrinseca dignità in tale momento. Arriviamo Arriviamo a questa formulazione con un po' di ritardo, ma ci arriviamo. Ci giungiamo dopo che il Comitato nazionale per la bioetica, nel lontano marzo del 2001, 2001, in un documento dal titolo «La terapia del dolore: orientamenti bioetici» dedicava un paragrafo *ad hoc* al tema del trattamento del dolore in travaglio di parto. Faccio mio quanto il documento riportava dicendo che il ricorrere alla sedazione del dolore del parto non si pone come alternativa al parto naturale, ma come mezzo che la medicina offre per compiere una libera scelta e per realizzare, con la sedazione del dolore, un maggior grado di consapevolezza e di partecipazione all'evento. Detta così, potremmo dire che è un'enunciazione

non solo a livello accademico), riscontriamo che con l'analgesia in travaglio di parto, oltre ad avere una maggiore *compliance* da parte della gestante stessa,

un diritto della partoriente scegliere un'anestesia che sia efficace e che dovrebbe essere inclusa tra quelle garantite, come dicevo nell'*incipit* del mio intervento, nei livelli essenziali di assistenza su tutto territorio nazionale.

dell'atto pratico in quanto anestesia loco-regionale - è che la dimensione della disarmonia che si incuneava nella sessualità, nella fecondità e nel rapporto generazionale (il fondamento di quella che viene definita l'immortalità della procreazione e della generazione) non era una condanna. Questo perché si andava a creare simbolicamente, attraverso la sofferenza, la dimensione propria dell'atto procreativo e generativo,

che non è una condanna, tanto meno qualcosa di auspicato o di auspicabile; piuttosto, essendo ontologicamente, intrinsecamente iscritto nella natura dell'essere umano, altrettanto è nella natura dell'essere umano trovare dell'essere umano trovare un antidoto, una soluzione, un intervento di ordine terapeutico alla sofferenza e al dolore, perché non sono una condanna, ma sono iscritti nella mortalità dell'essere persona. Il paradosso -

un mezzo, di un sistema per far sì che il dolore non ci sia o che venga attutito, c'è tutta la nobiltà sia dell'assistenza medica ed ostetrica, ma anche tutta la nobiltà e la grande dignità della procreazione e della generatività.

Mi aiuta in tutto questo lo sviluppo del dibattito di questa mattina: interventi molto precisi, molto puntuali,

tutti gli interventi concordino su due questioni: una di merito e l'altra di metodo. Il merito è che comunque le materie

La questione più di metodo, ma di grande significato: da tutte le parti è stato concorde il riconoscimento di uno sforzo di più culture, di più visioni dei problemi, di più appartenenze politiche certamente - siamo in Parlamento - ma tutte ragionevolmente confluite nel definire uno spazio di interesse comune, che poi sono gli interessi pubblici. La tutela della salute è un bene comune che va protetto, promosso, sostenuto; che va adeguato tempestivamente alle nuove esigenze che prepotentemente scendono in campo. Naturalmente esistono visioni diverse (aggiungerei: per fortuna). Anche stamattina, chiamandomi in causa, il senatore D'Anna ci ha riproposto le sue legittime visioni del problema:

Naturalmente, la materia è molto più complessa, e probabilmente nemmeno troppo pertinente, però vorrei dire semplicemente al senatore D'Anna che in ogni caso il nostro modello, con i suoi limiti e i suoi difetti (che nessuno ovviamente mette sotto al tappeto), è quello che meglio garantisce il rapporto tra la qualità delle prestazioni e l'investimento di risorse. Lì siamo in testa a tutte le classifiche. Il nostro modello è quello che, con il 6,8 per cento di spesa pubblica rispetto al PIL garantisce queste prestazioni.

Il nostro Servizio sanitario è quello che garantisce che entrino nelle disponibilità di tutti i cittadini, indipendentemente dalla carta di credito, le grandi innovazioni delle tecnologie, dei farmaci; e qualche volta in questi anni ho pensato come sarebbe stato diverso e più drammatico il peso della crisi se non avessimo avuto la sanità pubblica e la scuola pubblica. Si può anche non andare a cena, non cambiare la macchina, non andare al cinema, ma non si può non mandare i figli a scuola; non ci si può non curare.

questa legittima sollecitazione al dialogo in realtà non prefiguri una condizione per la quale concorrenza, mercato e sanità siano cose e fattispecie molto particolari e che l'unico modello di riferimento sia l'America dove la spesa sanitaria costituisce il

la forza innovatrice di questa novella, che non è una delega, sta proprio nel ridisegnare la *mission*, le funzioni e i ruoli, che sono diversi e profondamente modificati dallo sviluppo della sanità e della medicina. Se non li cambiamo e li rendiamo adeguati a reggere queste sfide, non avranno la capacità di assolvere quel ruolo di *governance* della complessità delle attività professionali sanitarie nella moderna sanità. È questa la forza innovatrice. Ho sentito poi obiezioni sul funzionamento e sulle elezioni. In realtà, alcune

che dovrà emanare il Ministero della salute: lì si potranno rivedere i bilanciamenti tra rappresentanza, rappresentatività, democrazia, durata delle cariche e così via. Mi pare inoltre non più rinviabile un ragionamento serio sulla sperimentazione e la ricerca clinica. Guardate, la ricerca e la sperimentazione sono le gambe su cui cammina il futuro il futuro della medicina come scienza (e non solo della medicina). O davvero siamo in grado di salvaguardarne l'integrità, di proteggerne e di promuoverne lo sviluppo pieno, oppure ci disegniamo un futuro asfittico. Credo che il provvedimento da questo punto di vista uno sforzo lo faccia.

e consegnare alla *Gazzetta Ufficiale* questo provvedimento, avremo sicuramente dato un contributo rilevante. Poi naturalmente si scontano, come spesso succede, obiezioni, critiche, opposizioni, visioni diverse, insoddisfazioni, ma è normale, perché è una materia complicata e difficile. Intanto questo è un buon passo, facciamolo decisi e convinti. *(Applausi

come sempre in questi casi, si dovrebbe ricominciare, perché pian piano i colleghi si sono resi conto dell'importanza di questo provvedimento, probabilmente sfuggita per modalità un po' tumultuose dei lavori dell'Aula. In Commissione abbiamo approfondito moltissimo e abbiamo fatto moltissime audizioni. Sono 1.200.000 i professionisti della sanità che stanno attendendo questo provvedimento.

insoddisfacente. Non c'è dubbio che sia così perché tutti avremmo voluto poter fare di più, ma questo è il punto di equilibrio. L'Unione europea stabilisce che gli ordini professionali in campo sanitario siano indispensabili per l'abusivismo professionale. La medicina transfrontaliera ci dice che dobbiamo entrare in Europa a testa alta con le professioni sanitarie riconosciute. L'abusivismo professionale non è un problema soltanto dei professionisti, ma innanzitutto di sicurezza dei cittadini. Esiste una dignità professionale per tutti, dai medici fino a tutte le professioni sanitarie che oggi riconosciamo. Questa

i percorsi formativi perché sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero della salute. Credo che, se ognuno facesse seriamente e bene la sua parte (Parlamento, Governo

Tuttavia, il punto di equilibrio che abbiamo raggiunto vuole che ci sia per tali professioni una "scatola", quella dei tecnici di radiologia, in cui, per la prima volta nella storia italiana, saranno obbligatoriamente previsti gli albi di queste professioni sanitarie. Questo è fondamentale. Abbiamo poi naturalmente medici, farmacisti infermieri, ostetrici, psicologi e biologi che avranno un ordine a sé. Ma se tocchiamo quella struttura che abbiamo previsto, oggi già molto complessa e quasi sperimentale, andiamo a rompere un equilibrio molto delicato. Penso dunque che la cosa dunque che la cosa più importante sia far uscire il provvedimento da quest'Aula, perché è fermo qui da troppi anni, e farlo approdare per la seconda lettura alla Camera, in cui, in accordo con i Ministeri, si potranno fare dei ragionamenti.

sono consapevole che ci sono contrarietà; sono consapevole che c'è una professione in particolare che è contraria all'istituzione di un albo composito di tecnici della riabilitazione,

e che, quindi, io accetto tutte le critiche mosse a me e al lavoro della Commissione e mi prendo le responsabilità che mi competono, come se le prenderà il Governo. Però, care colleghe e cari colleghi, mi volete dire cosa c'entra il dissenso con l'insulto, la minaccia e il dare dei ladri a tutti noi - perché questo è accaduto - in nome di una professione che dovrebbe, viceversa, curare in modo dolce le persone? Voglio essere chiara su questo punto, Presidente. Non è accettabile che vi sia una sovrapposizione che diventa conflitto di interesse etico nei confronti del Parlamento. Non si accetta; siamo persone perbene. Abbiamo lavorato unitariamente. Il dissenso è fisiologico, ma l'insulto, quando travalica, diventerà oggetto

di grandi disegni infiniti che poi non trovano applicazione: bisogna scegliere le priorità, e le priorità sono state la ricerca, che è fondamentale nel nostro Paese (la ricerca clinica e poi quella sui farmaci in particolare) e, in secondo luogo, la maternità, la maternità, perché prima di ragionare sui programmi di fertilità noi dobbiamo ragionare sulla sicurezza della maternità. Troppe donne, infatti, muoiono ancora oggi di parto, perché non vi sono i registri; perché ci sono Regioni dove i parti cesarei arrivano fino al 92 per cento, ed è uno scandalo e una vergogna di questo Paese! Quindi, noi dobbiamo andare verso

nell'articolo 1 c'è scritto esattamente quanto poi è presente nella legge Delrio. La fotografia degli ordini sta sulla fotografia del territorio delle Province, come nella legge del 2012. Tutto ovviamente si può migliorare, ma

non è la medicina delle donne. Voglio essere molto chiara al riguardo. Smettiamo di pensare che, come mi ha detto una sera una signora, adesso abbiamo anche l'aspirina rosa. La medicina di genere non è questa sciocchezza. La medicina di genere non è fatta per le donne; è fatta per corpi diversi ed elementi diversi tra uomini e donne, affinché non ci sia invasività dei farmaci sui corpi femminili, perché ci sia il rispetto degli uomini e delle donne e del loro sacrosanto diritto a venire curati. Non è quindi una quota, ma è un approccio metodologico e scientifico scientifico che ha grandissimo valore e in questo senso dobbiamo andare avanti. Tutto può essere fatto meglio. Ci rendiamo conto delle nostre insufficienze,

Non possiamo permetterci, ancora una volta, di voltare la testa dall'altra parte per piccole o grandi miserie quotidiane o per piccoli o grandi conflitti d'interesse. Siamo consapevoli che stiamo compiendo un passo molto più importante di quanto molti di noi possano pensare in favore di una migliore sanità e di un migliore Servizio sanitario nazionale.

qualche breve e spero utile osservazione a conclusione di questo che considero, senza infingimenti, un ottimo dibattito. Arriva in Aula un testo che - come è stato segnalato - è frutto di un lavoro molto intenso e anche molto proficuo

delle questioni ha sempre superato - in questa circostanza direi virtuosamente - posizionamenti di parte che spesso rendono il nostro lavoro non semplice, né in alcuni casi comprensibile. Si è determinato in Commissione un lavoro molto costruttivo, sicuramente grazie a chi presiede la Commissione, la presidente De Biasi,

che ha consentito un lavoro lungo e sicuramente datato, com'è stato fatto notare, perché molti degli elementi del disegno di legge facevano parte di attività parlamentari precedenti a questa legislatura e, quindi, c'è una sedimentazione complessa con la quale abbiamo dovuto fare i conti. È stato già detto, e vorrei ancora sottolinearlo, come in tema di sperimentazione dei medicinali a uso umano il provvedimento si spinga molto in avanti - questa è l'opinione del Governo spinga in avanti anche il nostro Paese, anche con delle specificità che sono state segnalate, soprattutto sulla medicina di genere, collocandolo finalmente in una prospettiva sempre più europea, dove i principi sulla sperimentazione scientifica, come quelli della semplificazione (risvolti anche economici a questa attività, ma soprattutto - mi sentirei di dire - assistenziali della ricerca e della sperimentazione), troveranno una più forte definizione che consentirà sicuramente al nostro sistema sanitario di cogliere meglio le straordinarie opportunità che, a livello mondiale, l'innovazione e la ricerca stanno portando avanti tumultuosamente. Vorrei segnalare solo

e del parto. Finalmente quel provvedimento è alle battute finali. Da qui a qualche giorno, dopo un lungo e faticoso lavoro delle Regioni, del Ministero dell'economia e dello stesso Ministero della salute,

È palese che una parte sostanziale del provvedimento è costituita proprio dalle innovazioni introdotte nel complesso settore degli ordini delle professioni sanitarie dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, che interviene con una riforma organica degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie al fine di rendere il nostro sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne una funzionalità nell'interesse prioritario dei cittadini.

La prima novità è rappresentata dalla definizione della natura giuridica degli ordini quali enti pubblici non economici e organi sussidiari dello Stato che hanno lo scopo di tutelare interessi pubblici connessi all'attività e all'esercizio dell'attività professionale. saranno enti dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Inoltre, viene chiarito in maniera netta di enti finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza pertanto gravare sulla finanza pubblica.

indicato come problema - che nell'individuare i compiti degli ordini medesimi, la pubblicità degli atti e degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti, il disegno di legge in che essi devono operare garantendo il rispetto di principi fondamentali quali l'accessibilità e la trasparenza, richiamandosi specificamente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla trasparenza nella pubblica amministrazione.

prevede una separazione netta tra funzioni istruttorie e funzione giudicante. A tal fine, in ogni Regione saranno costituiti appositi uffici istruttori di albo cui partecipa, oltre agli iscritti all'uopo sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime nominato dal Ministero della salute. Questi uffici istruttori, sulla base di esposti e su richiesta del Presidente della commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento e l'apertura di un procedimento disciplinare.

sanitari di radiologia medica e delle cosiddette professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. Le procedure per l'individuazione di queste professioni erano abbastanza note e sono convinto che il disegno di legge che stiamo per approvare chiarisca finalmente il quadro di questa organizzazione di ordini, albi e federazioni nazionali. Altra significativa novità è quella dell'istituzione dell'osteopata e del chiropratico. Per alcune di queste professioni

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la destinazione dei beni immobili confiscati all'autore del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria al sanitaria al patrimonio del Comune dove l'immobile è sito e la sua destinazione per finalità sociali e assistenziali.

reati ai danni delle persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali. Purtroppo la cronaca quotidiana ci segnala

che il conseguimento di più lauree o diplomi dia diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie presso le farmacie, ad eccezione, ovviamente, dei professionisti abilitati alla prescrizione dei medicinali,

la Presidenza, anche in considerazione dei criteri adottati nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 2.202, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 7.201, 8.0.200 e 11.0.200, nonché l'ordine del giorno G1.100 per estraneità al contenuto del disegno di legge in esame. Dichiara altresì inammissibile l'emendamento 3.216, in quanto privo del requisito essenziale della previsione dei principi e criteri direttivi per il conferimento della delega legislativa.

a sottolineare l'importanza di prevedere anche metodi alternativi, che rappresentino una concreta speranza per il futuro di non utilizzare gli animali nella ricerca, almeno per quanto riguarda la ricerca applicata. L'alternativa si fonda sul sistema delle tre R, *replacement, reduction and refinement*, ovvero sostituzione, riduzione e perfezionamento. di un percorso che coniuga l'interesse economico a ridurre i costi della ricerca, rendendola più efficace, produttiva e pertinente, con quello più specificamente etico di evitare il sacrificio degli animali in nome del progresso scientifico, quando ciò non apporta nulla di nuovo. In tutto il mondo si guarda con attenzione e speranza allo sviluppo di questi metodi di ricerca. Una forte accelerazione è stata impressa recentemente dalla nuova direzione dello European center for the validation of alternative methods, istituto tecnico della Commissione europea con il compito di studiare, promuovere e validare i procedimenti in cui non si fa impiego di animali. In ogni Paese membro dell'Unione europea hanno preso corpo valide iniziative, come l'European consensus platform for alternatives (ECOPA), a cui partecipano industrie farmaceutiche, enti governativi, istituti di ricerca e associazioni animaliste. Risulta fondamentale percorrere la strada dei metodi alternativi che, al di là delle questioni etiche, stanno diventando a livello internazionale una realtà di progresso scientifico. Mi permetto di fare un'altra considerazione. Questa mattina tutti hanno sottolineato il discorso della medicina personalizzata, della medicina di genere, di distinguere la ricerca anche per fasce d'età (adulto-bambino, razza, tipologia), perché sempre di più la ricerca avanzata si concentra addirittura sull'isotipo, sulla cellula specifica, sulla differenza di metabolismo. Quindi, sempre più, un certo modo di fare ricerca rimane antiquato, fuori dai tempi; ci sono altre tecniche e altre possibilità. Con questo emendamento si invita a individuare le modalità per promuovere questi

vanno avanti, la loro ricerca è apprezzata e garantiscono assunzioni e aumento del Prodotto interno lordo, per quanto riguarda il settore farmaceutico. Ampliare e investire in questo settore,

L'ordine del giorno G1.101 intende rafforzare l'impegno, già assunto dal Governo, nell'ambito della medicina di genere, in particolare attraverso il formale riconoscimento a livello nazionale di tale approccio e il sostegno alla ricerca sulla medicina di genere, anche incentivando la creazione, all'interno delle strutture sanitarie nazionali, di poli specificamente dedicati alla presa in carico dei pazienti di genere femminile. Ricordo che lo scorso 22 aprile è stata la prima giornata nazionale della salute della donna e in quella occasione vi è stato il manifesto della salute della donna in cui si è segnalata, in particolare, l'importanza della medicina di genere. L'ordine del giorno G1.102 mira a rendere il sistema di tariffazione delle strutture residenziali e semiresidenziali più equo e rispondente ai reali bisogni della popolazione,

un provvedimento su cui questa mattina ho sentito la Commissione autocomplimentarsi. Questo fa piacere, perché vuole dire che lavorare con passione, coinvolgimento e motivazione è una cosa positiva;

fine, l'intero provvedimento è una serie di titoli che dovranno avere esplicazione dettagliata e potrebbero anche riservare delle sorprese. Ciò premesso, con questo emendamento si prevede soltanto di individuare individuare delle modalità per la promozione di una sperimentazione con metodi alternativi a quello animale. È quasi un ordine del giorno,

questo emendamento è molto importante perché mira a regolare il finanziamento privato ai progetti di ricerca in modo da restringere le possibilità di alterazione dei risultati per ragioni di interesse particolare. In particolare, per i progetti riguardanti la ricerca epidemiologica ambientale e la valutazione degli effetti sulla salute, si chiede di adottare precisi protocolli conformi al documento dell'International society for

Orellana che nella legge di stabilità di quest'anno il meccanismo di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stato costruito in maniera più fluida e veloce, perché c'è una Commissione che paradossalmente potrebbe aggiornarli anche prima dei due anni, se ci fosse una necessità e un'evidenza

riforme, di razionalizzazione e soprattutto di utilizzo di metodi telematici per cui a livello centrale possiamo avere l'elenco di tutti gli appartenenti agli albi e agli ordini, non non si capisce perché non si eliminino gli ordini provinciali e si mantengano quelli regionali. Io credo che un ordine regionale sia più che sufficiente, soprattutto nell'ottica dell'eliminazione delle Province.

i decreti attuativi e i decreti delegati si preoccuperanno soprattutto di rendere più democratica la votazione all'interno degli ordini, ritiro gli emendamenti 3.207, 3.208

semplicemente per specificare che l'equipollenza dei titoli validi per l'iscrizione a un albo professionale debba riguardare anche quelli conseguiti all'estero.

«Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive». Per l'esercizio dell'attività sanitaria di cui al presente comma è necessario il possesso della laurea in scienze delle attività motorie e sportive

o che servono - dopo che il fisioterapista ha effettuato le manovre di riabilitazione - a mantenere il mio stato fisico pretendo che quella persona sia iscritta ad un albo, dove io posso accertare che si tratta di un laureato in scienze motorie. Vi posso garantire che pochi

numero di telefono e indirizzo, avrebbe potuto venire da me. Voglio anche aggiungere che sono uno di quei medici che ha molto piacere che si sia cominciato a capire che chiropratico, osteopata, fisioterapista, psicologo, medico debbano non collaborare ma lavorare insieme, perché ci sono tanti percorsi, rispetto ai quali ciascuno deve essere in grado di svolgere la sua parte, senza la paura

Ho sostenuto apertamente la formazione di un albo di osteopata e chiropratico. Mi si dice che tutto questo non può essere fatto perché abbiamo un equilibrio della struttura. Non capisco francamente dove si rompa questo equilibrio. Se ho persone laureate in scienze motorie,

chi mette le mani sul paziente o fa qualcosa che si rivolge alla salute del paziente, deve essere iscritto ad un albo, e non è un caso che scienze motorie sia inserita nella facoltà di medicina e chirurgia.

Ho espresso alla senatrice De Biasi il mio rammarico per tutte le persone che in maniera volgare difendono una fettina del loro guadagno. mi dissocio perché non sono mai stato uno che in maniera volgare difende una fettina del proprio guadagno. Sono qui per difendere gli interessi del paziente, che in questo momento sono anche gli interessi di una piccola categoria.

ottenuto il riconoscimento in uno specifico ordine professionale. Credo che l'ordine del giorno di impegno al Governo ad adottare specifiche misure al fine di istituire nuovi Ordini professionali per quelle professioni sanitarie che superano i 20.000 iscritti agli albi sia un segno di apertura e disponibilità che pacifica il clima di tensione che si è creato. Inoltre, credo apra una porta ad istanze che vanno considerate come legittime, soprattutto in funzione di quelle figure ormai radicate nell'ambito del Sistema sanitario e che, giustamente, attendono attendono il conseguimento di questo traguardo, che penso non debba e non possa essere negato.

Credo sia importante che l'emendamento 3.228 possa trovare consenso, perché eviterebbe di incappare in malintese definizioni professionali, utilizzando termini termini propri delle professioni che qui vengono regolamentate, per individuare attività professionali diverse. Mi riferisco, per esempio, a un badante che può definirsi infermiere senza averne il titolo.

a produrre un metodo di semplificazione e una procedura di elezione e di costruzione sociale più moderna delle strutture e degli Ordini. vogliamo, in un provvedimento dove si vuole ammodernare la visione e renderla più conforme ai parametri europei, ancorarci a meccanismi vecchi, risulta necessario, a mio avviso, che ogni Ordine promuova un'adeguata pubblicità dei candidati, per renderli appunto riconoscibili agli iscritti che sono chiamati ad esprimersi, nonché un altro meccanismo, ovverosia proporre e suggerire l'espressione di un massimo di cinque

MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, forse è il caso che si attenda l'esodo In ogni caso, ho interesse a parlare per gli atti e per chi di dovere, ferma la gratitudine per chi resta. In data 17 maggio scorso abbiamo ricevuto una lettera dal Presidente del Senato che, per opportuna conoscenza, ci trasmette una lettera

di essere capofila per la formazione della posizione nazionale sull'accordo. Credo che dobbiamo dargli riconoscimento per questo ambito traguardo;

In realtà, la «massima trasparenza e diffusione» sono - basta leggere la modulistica - la massima realizzazione del segreto. alcuni punti. In primo luogo, la sala è vigilata dall'Arma dei carabinieri. In secondo luogo, ci sono due turni di quattro ore per tre giorni. Ogni senatore ha comunque diritto a un solo turno di un'ora. Il senatore deve dichiarare l'effettiva necessità di conoscere il testo, quindi si immagina che si possa voler trasmettere informazioni a una potenza straniera, oppure organizzare un un corteo anarchico o quant'altro. Il senatore deve dichiarare la sua personale responsabilità: forse si dimentica che è ancora vigente e non ancora riformato l'articolo 68 della Costituzione. *(Applausi dai Per tranquillità, segnalo che questa materia è comunque di competenza anche del nuovo Senato, perché in qualche modo ha a che vedere con l'appartenenza all'Unione È vietato, ovviamente, riprodurre il testo, è permesso prenderne nota a mano, ma è vietato che la nota contenga lo stesso testo del documento che viene offerto per la massima trasparenza e consultazione. Suggerirei anche che con il Ministro, se è disponibile, si sorteggi un articolo di quelli e ce lo spieghi: vedremo se sarà capace di farlo, dato il carattere molto criptico di quei testi. In conclusione, rispetto la posizione degli Stati Uniti d'America, ho molte difficoltà a rispettare la posizione europea e nazionale. C'è stata una fase nella storia in cui i trattati sono stati segreti e quella è una fase che ha portato ad esiti tragici a ridosso della Grande Guerra. I trattati non possono essere segreti: può essere segreta la trattativa, ma non può essere segreto il testo dei trattati. *(Applausi dai Gruppi mezzo, ovvero è quasi segreto ed è quasi pubblico, attraverso una procedura che dimostra il dinamismo del signor Ministro, ma anche l'anacronismo storico e devo dire che in politica e tra gli Stati c'è una sola cosa che è temibile più di tutte: il ridicolo.

la ringrazio per avermi concesso la possibilità di aggiungere le mie parole a quelle ben più autorevoli del senatore Tremonti. Ci voleva un intervento autorevole come il suo, per provare a far registrare all'Assemblea l'imbarazzo che credo tutti abbiamo provato nel leggere ieri quella missiva, con le procedure così scritte, che sono senz'altro foriere come minimo di malintesi, quando non di tragedie annunciate.

presentare una mozione in Senato, affinché il Presidente del Senato si faccia rappresentante dei parlamentari, che pretendono di conoscere - non in quella formula, non con quelle modalità, ma con modalità ben più trasparenti - il contenuto vero di questo accordo. Ricordo benissimo la Commissaria europea quando, in occasione di un'audizione convocata dal presidente Chiti, si rammaricò per l'errore commesso dalla Commissione europea, che in quella fase rendeva disponibile il contenuto dalle trattative in corso sul TTIP guardi un po' - presso le sedi delle ambasciate americane nei Paese europei e non, ad esempio, presso la sede dell'Unione europea in ciascuno dei Paesi aderenti. Signora Presidente, sarà nostra cura,

mi unisco all'appello dei colleghi e sostanzio ancora di più questa richiesta, evidenziando altri punti importanti di questa direttiva per la consultazione, che ci è arrivata dal neoministro Calenda. il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 6 novembre 2015, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva» alla legge sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto». Vorrei ricordare a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando in questo momento - perché naturalmente non serve ricordarlo a voi, colleghi - che stiamo parlando di un accordo

Il Movimento 5 Stelle si sta battendo da anni contro questo trattato, che sarà distruttivo per la nostra economia. Riteniamo che le persone che hanno l'effettiva necessità di conoscere questo trattato e i contenuti del negoziato siano tutti i cittadini italiani.

lasciato tutti noi, senatori e parlamentari, a dir poco sgomenti. Vorrei precisare che la parte che sarebbe consultabile, in queste forme così è solo quella già approvata. Vi è ancora un'altra parte totalmente segreta a cui, come si vede, non possiamo accedere in alcun modo. Presidente, ora qui si pone un problema. Il TTIP riguarderà non solo l'economia del nostro Paese e gli interessi nazionali, ma anche la salute dei cittadini,

presentiamo lì e non obbediamo a tutte le prescrizioni che sono state indicate dal neoministro.

potrebbe avere conseguenze molto gravi, non solo per l'impatto sull'articolo 68 della Costituzione, ma davvero e sostanzialmente sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

collega De Petris. Penso che il Presidente del Senato e la Presidente della Camera debbano approfondire quali sono i diritti dei parlamentari nel nostro Paese in rapporto agli atti di Governo, punto e basta.

Di incondizionato nei rapporti tra Stati c'è solo la resa quando si perde una guerra; forse ne abbiamo persa qualcuna senza saperlo. È doveroso che ci sia trasparenza su cosa ha determinato la resa incondizionata della nostra Repubblica. *(Applausi dai Gruppi Signora Presidente, credo che sia opportuno che il Senato e la Camera facciano le loro valutazioni rispetto alla questione che è stata così compiutamente esposta dal senatore Tremonti. Vorrei indurre due riflessioni.

Nella fattispecie, siamo nel corso di una trattativa in cui ci sono delle parti di Trattato che non sono compiute, quindi siamo in una condizione che è di di Trattato non compiuto e non definitivamente definito e con una trattativa che è in corso e che richiede delicatezza nell'informazione.

Purtuttavia, siamo di fronte ad una modalità che rende per il Parlamento agibile e conoscibile il Trattato nella sua struttura attuale e che mette il Parlamento nella condizione di chiedere al Governo, in qualunque momento, chiarimenti attraverso le procedure classiche di dialogo tra Governo e Parlamento. In tutti i casi, se il Presidente del Senato e la Presidente della Camera vorranno avere un'attenzione particolare alle modalità piuttosto che al contenuto del Trattato (perché sul contenuto del Trattato facciamo una discussione di natura politica e non metodologica), da parte nostra non vi sarebbe nessun tipo di resistenza. Sarei per dire che un atteggiamento ponderato e ragionevole

Signora Presidente, mi permetto di far notare al collega Sangalli che la prudenza che lui chiede dovrebbe portare il Governo ad evitare giudizi definitivi, perché se è vero che siamo in una situazione provvisoria per cui c'è bisogno di tutte queste attenzioni, dare giudizi definitivi e in qualche modo compiuti, contraddice evidentemente le ragioni di prudenza che si pongono. quando c'è una situazione di questo tipo, non si rende difficile la consultazione, non ci si ferma a metà del guado, non si dice «è segreto ma è pubblico, anzi è un poco pubblico e un poco segreto e se riuscite a non capirci niente è tanto meglio». In questi casi, evidentemente, c'è uno strumento diretto, al quale il senatore Sangalli stesso ha fatto riferimento, e cioè credo vi siano tutti gli estremi affinché il Senato chiami

dire alcune cose e tacerne altre, ma questo è un procedimento chiaro. Quello che è stato adottato, francamente, è non soltanto opaco, ma addirittura ridicolo. il Gruppo della Lega Nord non può che essere assolutamente concorde sulla necessità che il Ministro degli affari esteri venga in Aula e riferisca in merito a questa situazione. La missiva che abbiamo ricevuto è firmata dal neo ministro Calenda, ma qui certamente, come è già stato ribadito, si tratta di affari esteri e per di più con modalità che non tengono conto non dico della semplice dignità, ma del ruolo di rappresentanti democraticamente eletti dal popolo, dei parlamentari. Qui dentro noi non abbiamo desiderio di conoscere le carte per sfizio o per cronaca, ma per giusta relazione nei confronti dei cittadini. Negare o limitare l'accesso agli atti è una pratica incostituzionale, perché vorrei vedere che cosa accadrebbe nel momento in cui qualsiasi parlamentare, in quest'Aula, rivelasse quei documenti. Sarebbe un atto di pura democrazia, così come sarebbe un atto di pura oppressione del diritto democratico se questo venisse impedito. Signora Presidente, ribadisco il concetto: il Ministro degli affari esteri venga in Aula e riferisca con urgenza in merito a queste modalità, quantomeno quantomeno bizzarre, di consultazione. Riteniamo che il Governo debba mettere totalmente a disposizione del Parlamento e dei cittadini questa documentazione, non accorgendosi peraltro di un paradosso, cioè che le carte sono già state pubblicamente rese note, anche sulla stampa, nei giorni scorsi. Quindi limitare ulteriormente vuol dire mettere una toppa che è molto peggiore rispetto a quello che evidentemente il ministro Calenda voleva scrivere nella sua missiva.

Io mi trovo da un mese in questa condizione, perché, avendo visionato le carte di trentasei anni fa, relative al maggio‑giugno 1980 (Ustica e Bologna), conoscendone i contenuti ed avendoli potuti annotare,

Lo dico perché non si può essere accusati di essere dei depistatori, come ogni giorno leggo pubblicamente da Bologna. Le carte vengono tenute coperte e non si può fare un confronto con l'opinione pubblica su chi è veramente il depistatore. In questo caso si possono andare a vedere, ma non si può fare un dibattito,

le parole «libertà», «democrazia» e «trasparenza» sono tutti concetti eterei, indefiniti, persino ambigui, laddove non trovino corrispondenza con principi, norme, limiti, regole e procedure capaci di dar loro un corpo, una coerenza, un universo simbolico di riferimento. Non sarebbe questa un'Aula di un Parlamento di uno Stato democratico, se non ci fosse un Regolamento da rispettare, ispirato a principi democratici. Non può esistere un'organizzazione che pretenda di essere democratica e che non sia regolata secondo norme coerenti con i principi democratici. Ciò che è successo recentemente al sindaco di Parma Federico Pizzarotti, persona onesta e coerente, è solo l'ennesimo esempio di come la seconda forza politica del Paese utilizzi a sproposito parole nobili come «trasparenza» e sia dedita invece a colpire ogni voce interna capace di pensiero critico o dialettico, arrivando ad inventarsi regole o procedure *contra personam*, pur di far fuori chi non si allinea. Il Movimento, nato per promuovere la democrazia dal basso, è diventato il partito del bispensiero, ossia di quel meccanismo psicologico, descritto da Orwell, che consente di sostenere un'idea e il suo opposto, in modo da non trovarsi mai al di fuori dell'ortodossia. Per cui si può credere di promuovere la democrazia dal basso, facendosi comandare e dirigere da una o due persone (anche per dinastia). Pizzarotti è la testimonianza del Movimento come doveva essere, per come era nato. Per questo motivo era da tempo giunto il momento di eliminare politicamente, isolare, nascondere, cancellare, delegittimare Pizzarotti e abbandonarlo all'oblio. Voi parlamentari - che ovviamente non ci sono, perché vogliono lavorare dal lunedì al venerdì, ma poi, quando ci sono i giorni convenuti, in Aula non ci sono, ma vanno via veloci veloci come cavallette - in tutti i casi, del Movimento 5 Stelle vi eravate illusi, con l'annuncio del passo indietro di Grillo. Prendetene atto, però: con l'attacco a Pizzarotti muore definitivamente nel vostro partito l'idea di voi stessi,

La seduta è tolta